Grazie

nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunico che in data 16 maggio 2016 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno* «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza» (2389).

europeo, italiano e sardo, Pinuccio Sciola. Dice di lui Beppe Severgnini: «Pinuccio Sciola era un uomo roccioso. O una roccia antropomorfa, fate voi. Aveva gambe solide, braccia muscolose, mani robuste, capelli forti, sguardo deciso. Non era piccolo: era conciso. Il riassunto della Sardegna. Ci sono artisti che somigliano alla propria terra, altri che potrebbero essere nati e cresciuti dovunque. Pinuccio Sciola era sardo fino all'ultima molecola». Lo scultore sardo è scomparso lo scorso 13 maggio a settantaquattro anni. Di lui, che ha dato lustro, come altri nati in Sardegna, all'Italia, si deve ricordare soprattutto la profonda sensibilità verso le radici dell'umanità, che affondano nella terra e si innervano nella roccia. La pietra, attraverso la sua imponente opera, non solo si anima nella figura, ma parla con la più naturale delle musiche, ognuna con suoni diversi. Le pietre di Sciola, scolpite con fessure profonde, sono impiantate nel mondo intero, dal suo San Sperate, il paese dei *murales*, all'Argentina, a Tokyo, al Giardino della pace di Assisi, a Roma. Un grande sardo, artista di formazione europea, come dice di lui Arturo Quintavalle, le cui opere attraversano il mondo pur avendo scelto lui di non essere un artista sul mercato. A lui va il nostro ricordo, la nostra gratitudine, il nostro omaggio: *ariosu*, Pinuccio.

31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare*** *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato già approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previe dichiarazioni di voto. Avverto altresì che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, in seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale sarà approvato se nella votazione finale otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Il relatore, senatore Russo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima deliberazione presso i due rami del Parlamento, è stato definito dalla Commissione affari costituzionali dopo un ampio esame, a partire da due proposte, la prima di iniziativa del senatore Pegorer, la seconda di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Siamo, quindi, chiamati in seconda deliberazione a pronunciarci in via definitiva sul provvedimento, senza possibilità, com'è noto, di apportare modifiche o avanzare proposte di stralcio. L'oggetto del disegno di legge - mi preme sottolinearlo e ricordarlo all'Assemblea - è la modifica dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale, con l'obiettivo di sopprimere le Province, adeguando l'ordinamento della Regione al processo di riforma istituzionale, mirando, tra l'altro, a semplificare il sistema degli enti locali. In secondo luogo, il disegno di legge punta a permettere l'istituzione delle Città metropolitane, caso in evidente consonanza con quanto previsto a livello nazionale. Il testo reca, poi, altre disposizioni che brevemente provo a riassumere. Anzitutto, il primo articolo, aggiunto proprio nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, modifica il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto, che definisce il territorio regionale, al fine di adeguarlo alle modifiche amministrative intervenute nel corso del tempo. Nel nuovo testo, infatti, si specifica che «La Regione comprende il territorio delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste». L'articolo 2 modifica, invece, l'articolo 7 dello Statuto in materia di potestà legislativa della Regione, stabilendo che la Regione possa istituire, con nuove leggi, Comuni anche nella forma di Città metropolitana. Il nuovo articolo 10 dello Statuto, come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge, prevede poi che lo Stato possa delegare con legge l'esercizio di proprie funzioni amministrative anche alle Città metropolitane. L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 dello Statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della Regione. La disposizione sopprime il termine «Province», inserisce il richiamo all'ente Città metropolitana e adegua il testo ai principi dell'articolo 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà. L'articolo 5 modifica il secondo comma dell'articolo 15 dello Statuto, concernente l'elettorato passivo per le elezioni del Consiglio regionale, al fine di abbassare l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo da 25 anni, come nel testo vigente, alla maggiore età. L'articolo 6, nel modificare l'articolo 27 dello Statuto, concernente l'iniziativa legislativa, diminuisce il numero di firme necessarie per la presentazione di un progetto di legge regionale da 15.000 a 5.000. Gli articoli 7, 8 e 10 modificano rispettivamente gli articoli 51, 54 e 62 dello Statuto al fine di comprendere, nella nuova definizione del complesso degli enti locali della Regione, anche i Comuni nella forma di Città metropolitane. Gli ambiti d'intervento sono i seguenti: l'articolo 51 dello Statuto concerne le entrate della Regione e la possibilità di istituire tributi propri, l'articolo 54 prevede la possibilità per la Regione di assegnare agli enti locali una quota delle entrate regionali, mentre l'articolo 62 riguarda riguarda le funzioni del Commissario di Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia. L'articolo 9 sostituisce l'articolo 59 dello Statuto, stabilendo che sono i Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, la base dell'ordinamento degli enti locali della Regione. Essi sono enti automi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto. L'articolo 11, che novella l'articolo 66 dello Statuto, consente alla Regione di decentrare i propri uffici nel circondario corrispondente alla giurisdizione del tribunale di Pordenone per le funzioni amministrative. Infine, l'articolo 12, recante disposizioni transitorie, stabilisce la soppressione delle Province della Regione Friuli-Venezia Giulia esistenti, a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e comunque non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. Con la medesima legge regionale sarà disciplinato il trasferimento delle funzioni delle Province ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane o alla Regione, nonché alla conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite e la successione nei rapporti giuridici. Al comma 3 si prevede che fino alla loro soppressione, le Province saranno disciplinate dalla normativa previgente. soltanto qualche giorno fa, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Udine, è stato celebrato il 40o anniversario del terribile terremoto che sconvolse il Friuli, è stato ricordato dal nostro Presidente della Repubblica non solo come un esempio della straordinaria capacità delle genti friulane di reagire ad una calamità terribile, ma anche per la straordinaria esperienza amministrativa che permise alla Regione Friuli-Venezia Giulia e ai Comuni interessati dal sisma di dare una risposta straordinaria, che ha portato alla ricostruzione

ove attuata e valorizzata, la specialità diventa un arricchimento ed un modello possibile per il

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia al nostro esame, di particolare importanza e complessità, si prefigge obiettivi ambiziosi: garantire una puntuale realizzazione della legge Delrio e, al contempo, ridefinire in modo ordinato e sistematico la razionalizzazione dei livelli di governo territoriale, tenendo ben presente le specificità locali, come appunto la Regione Friuli-Venezia Giulia. Il dibattito politico avvenuto in Friuli-Venezia Giulia nel corso dell'*iter* ha sollevato diversi temi non più demandabili: il ruolo delle Città metropolitane e di tutti gli altri livelli di governo territoriale, nonché il valore delle autonomie, per quanto attiene alla gestione delle istanze politiche primarie del territorio. Non a caso, già la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 ha costituito un primo provvedimento legislativo di riordino del sistema alle autonomie locali, il quale è intervenuto a distanza di dodici anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1993, che ha attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia una potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Siamo quindi oggi chiamati ad interagire, in qualità di Assemblea del Senato, con tale iniziativa legislativa. È importante che Parlamento e Regione si confrontino sui temi autonomisti, con l'esito di integrare il dibattito locale e quello parlamentare in modo sinergico. Senza dubbio la forza propulsiva della predetta legge è stata quella di configurare gli enti di secondo livello come strettamente legati da un rapporto di interdipendenza politico-funzionale con i Comuni e con le rispettive circoscrizioni territoriali. Ho premesso ciò perché oggi, con la presente discussione, non solo contribuiamo ad un percorso già tracciato, che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale, ma affrontiamo anche la singolarità del territorio con un'attitudine autonomista, che ha negli anni ottenuto la specificità in considerazione proprio della diversità che rappresenta al suo interno. In particolare, da tener ben presente è il perno attorno a cui ruota il rinnovato disegno istituzionale, che è il principio di sussidiarietà, così come sancito nell'articolo 118 della Costituzione, nonché lo stesso significato autonomistico voluto dalla riforma del 2001, che si è poi evoluto alla luce della giurisprudenza costituzionale. Ed è proprio il suo *status*, peculiare e prossimo alle istanze del territorio, a garantire - in un'ottica futura, ma ormai sempre più concreta - un accesso facilitato e puntuale, acquisendo nuove competenze e tutelando tipicità territoriali e minoranze linguistiche. Il mio invito, quindi, è di concentrarsi sulla bontà e la lungimiranza politica degli obiettivi che il provvedimento si pone, in un quadro di per sé complesso, caratterizzato da una pluralità di interventi normativi realizzati in un ristretto contesto temporale. Occorre dare atto che già nei precedenti passaggi parlamentari si è svolto un buon lavoro, essendo consapevoli che difficilmente si poteva fare di più, considerato il vigente quadro di riferimento costituzionale in materia di autonomie A tal proposito, mi permetto di rilevare che, all'articolo 4, comma 2, del presente provvedimento, si prevede anche l'obbligatorietà di esercizio associato delle funzioni comunali. Quindi sarà la stessa Regione che dovrà trovare una soluzione di accordo con i vari Comuni facenti parti del nuovo livello ordinamentale come le UTI, oggetto di più osservazioni da parte di svariati Comuni della Regione. Inoltre, desidero far presente che le modifiche contenute all'articolo 6 riducono da 15.000 a 5.000 il numero degli elettori firmatari di iniziative per la formazione delle leggi regionali. Nello specifico, gli emendamenti proposti dal sottoscritto e dal relatore e presentati in prima lettura rimarcano la volontà politica già manifestata dalla legge regionale del 2006; quindi definitivamente la Città metropolitana come elemento in grado di valorizzare le potenzialità economiche, tecnologiche, culturali e sociali del territorio interessato, intervenendo sullo sviluppo economico e sui flussi di merci e persone, nonché sulla pianificazione territoriale. Rimarrà quindi facoltà del territorio adeguarsi eventualmente in questa direzione. La modifica dello Statuto regionale è stato un momento di interessante interessante raffronto e di analisi, che ha portato tutti noi a comprendere meglio le dinamiche legislative della Regione, in considerazione anche delle rispettive funzioni con il Parlamento. *(PD)*. Signor Presidente, illustri colleghi, oggi non ci accingiamo solamente a decidere del futuro di un intero territorio, ma stiamo per scrivere una nuova pagina della storia istituzionale italiana. Con l'approvazione delle modifiche allo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia stiamo operando un cambiamento epocale all'interno dell'assetto istituzionale italiano. Il processo di riforma che sta ora investendo la mia Regione potrebbe, fra pochissimo tempo, manifestarsi anche nel resto del Paese, pertanto asserisco senza difficoltà alcuna che, in questo storico momento, il Friuli-Venezia Giulia è un precursore dei tempi. Con la rimozione delle Province dallo Statuto, la Regione si sta ponendo all'avanguardia nel riassetto istituzionale italiano, soprattutto se si considera che, con la definitiva realizzazione della riforma del Titolo V della Costituzione, le Province non saranno più previste anche nel resto del Paese. Bisogna premettere che in Friuli-Venezia Giulia si è già iniziato a superare le Province, con una riforma degli enti locali che rispetta i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza. una riforma che porterà ad una nuova organizzazione dell'assetto istituzionale regionale e al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini. Si tratta quindi di un processo complesso, che porterà ad un sistema integrato basato su due pilastri: la Regione e i Comuni.

di effettuare una complessiva riallocazione delle funzioni amministrative nella Regione. Queste Unioni eserciteranno in forma associata funzioni comunali e di area vasta, sia provinciali che regionali, dando quindi vita ad una nuova forma di governo del territorio, in grado di lavorare in maniera più efficiente a favore del cittadino. I Comuni saranno così tenuti ad operare insieme, generando tutta una serie di processi positivi, fra i quali lo scambio di buone pratiche e la specializzazione dei servizi. Quello che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha fatto con il rimodellamento della propria architettura istituzionale e la conseguente razionalizzazione delle autonomie locali è di fatto una delle massime espressioni di utilizzo della propria specialità. Il Friuli-Venezia Giulia sta quindi dimostrando un'autonomia seria, determinata e coerente, esercitando le proprie competenze per portare ad un efficientamento dei servizi e ad una migliore gestione del denaro pubblico. Il Friuli-Venezia importante di un cambiamento capace di migliorare la qualità della vita della popolazione ivi residente. Il testo che andremo a votare prevede anche la possibilità di istituire, come è stato detto, Città metropolitane nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Va ricordato che questo intervento modificativo è stato molto dibattuto e anche criticato dalle forze politiche nel Consiglio della succitata Regione io stessa lo trovo alquanto forzato, anche perché la Regione ha già iniziato un processo di profondo cambiamento che porterà i Comuni a lavorare insieme. La Città metropolitana rischierebbe dunque di sovrapporsi alle già costituite Unioni territoriali intercomunali. ribadito che non è previsto alcun obbligo di istituzione della Città metropolitana e che in forza della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, la disciplina in materia è demandata alla Regione. Bene, quindi, ma non possiamo concederci il lusso di perdere ulteriore tempo. Il Friuli-Venezia Giulia deve poter ragionare con serenità sul proprio futuro e portare a termine una riforma, che renderà più moderna ed efficiente l'organizzazione dei propri servizi locali. È tempo di scelte coraggiose, come quelle che sono state fatte da noi. Quella che ci prestiamo ad approvare è una buona legge ed è la stessa Regione autonoma ad aver chiesto di approvarla il prima possibile. Invito quindi i colleghi a liberarsi dagli indugi e mi esprimo a favore di questo disegno di legge, che permetterà ad un intero territorio di crescere, di progredire e di svilupparsi. Signor Presidente, innanzitutto forse avrei avuto il modo e il tempo di chiudere il mio intervento prima, se educatamente lei mi avesse permesso di avanzare le mie richieste, che andavano nel senso di invertire l'ordine del giorno.

che si chiama Sappada - lo sottolineo nuovamente - che da troppi anni attende una propria ridefinizione. Da parte nostra chiediamo fortemente che venga ripreso questo argomento.

questo passaggio, lo ripeto; anzi, è proprio un insulto a quello che è stato l'*iter* di una comunità, per la quale combatteremo, al di là di ogni scelta che verrà fatta.

Ci troviamo di fronte a una delle rare occasioni in cui uno Statuto di autonomia speciale viene sottoposto all'Assemblea del Senato e all'Assemblea della Camera per una sua modifica. In questo caso la modifica avviene perché la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia hanno inteso adeguare il proprio Statuto ad una riforma

È significativo che il Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia abbia assunto questa determinazione, perché significa essere coerenti con il processo di ridefinizione dell'architettura istituzionale

Va dato atto e merito al Consiglio del Friuli-Venezia Giulia di avere assunto con coraggio il tema del riordino istituzionale all'interno dei propri confini, di avere immaginato, in una realtà di 1,2 milioni di abitanti, che i livelli importanti politicamente rappresentativi - tutti i livelli delle autonomie locali sono importanti, ma intendo quelli politicamente rappresentativi - siano i Comuni L'ente intermedio, che è stato cambiato - non è più la Provincia ma saranno le Unioni territoriali intercomunali intercomunali - ha assecondato il disegno statale di semplificazione del quadro, senza con questo far venire meno quelli che sono i fondamenti Repubblica delle autonomie; anzi, producendo una valorizzazione delle autonomie comunali e, attraverso le loro unioni, dando una forma di governo che sia più direttamente a contatto con i cittadini con i cittadini e con le esigenze che i cittadini rappresentano. Questo è stato ed è un passaggio estremamente significativo ed è importante che la Camera e il Senato abbiano accolto questo sforzo riformatore di una Regione a Statuto speciale. È importante che questo sia accaduto; lo è per il Friuli-Venezia Giulia e per l'architettura istituzionale delle autonomie locali della nostra Repubblica. Per questo spero e mi auguro che questa sera il Senato possa dare il proprio definitivo voto favorevole a questa proposta di riforma.

che dalla legge Delrio in poi avete causato e state causando a questo Paese. Nello specifico, per quanto riguarda il Friuli è molto semplice: si vogliono cancellare le quattro Province per creare 17 Unioni di Comuni che di fatto diventeranno delle mini Province.

passeranno dagli attuali 45 milioni di euro a circa 65 milioni. E questo non lo dico io, non lo dice la Lega, ma la CGIA di Mestre. sentire questa sera, da parte del Sottosegretario o del relatore, un giudizio, un parere, anche una giustificazione davanti a questi dati che ritengo importanti. Magari si sono sbagliati, o magari abbiamo capito male noi, ma credo sia significativo questo passaggio, perché alla base della scelta, dal nostro punto di vista sconsiderata, della legge Delrio, per arrivare oggi allo Statuto del

un esempio: abbiamo visto e sappiamo per certo che la gestione delle strade passerà alla alla Regione in questo caso, e anche qui avremo un aumento di spesa - dicono - di 95 milioni di euro. Sono

che per noi è molto evidente: alla base di tutto non c'è assolutamente un calcolo, un disegno sereno e pulito per avere quello che avete dichiarato,

per accentrare tutto a Roma e nello Stato centrale. Questo è il disegno chiaro che noi leggiamo e che abbiamo letto in tutte le azioni fatte dal Governo.

quarant'anni fa in quella terra e che negli anni successivi ci ha consegnato un esempio di politica del territorio che resterà sempre nella storia.

ma se mai dovesse replicarsi per qualsiasi motivo un'emergenza simile, con quello che state creando sarà molto difficile, a prescindere dal DNA che contraddistingue la gente di quella terra, riuscire a replicare ciò che è stato fatto in Perché il sistema amministrativo che voi state compromettendo mette in forte discussione ogni azione sul territorio, e alla base c'è un disegno molto chiaro; lo state consegnando al Paese e lo stiamo vedendo con tutte le Province. Altro che risparmio:

ci sono già dei problemi, purtroppo. Sono Province che funzionavano. Abbiamo fatto gli amministratori ed io posso permettermi di dire, caro Bressa, di aver fatto l'amministratore in quella Provincia. Ma oggi posso constatare, dati alla mano, che non funziona più, funziona molto meno bene. Il futuro cosa ci riserverà? Non lo so. Sono certo di una cosa: c'è un futuro scritto per voi e lo leggeremo insieme il prossimo autunno, ad ottobre. Stia sereno.

questa proposta di legge ha principalmente l'obiettivo di sopprimere le Province e delineare un assetto istituzionale che contempli due livelli di Governo: la Regione e i Comuni. Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la proposta di legge costituzionale in modo da riorganizzare il sistema delle autonomie locali secondo il principio di sussidiarietà verticale, ma anche di adeguatezza. Infatti, è opportuno investire di maggiore responsabilità i Comuni, che sono i livelli istituzionali più vicini ai cittadini e che conoscono maggiormente le problematiche e i bisogni del territorio. Per la Regione Friuli-Venezia Giulia, quindi, occorre delineare un sistema più razionale che contempli due soli livelli di governo politico, espressione della sovranità popolare, cioè la Regione e i Comuni. La proposta di modifica dello Statuto va, infatti, necessariamente letta assieme alla riforma dell'ordinamento degli enti locali, portata avanti dalla Giunta regionale friulana, ovvero la cosiddetta riforma delle unità territoriali intercomunali. Con la riforma costituzionale che ci apprestiamo a votare, il Parlamento discute l'abrogazione delle quattro Province, mentre nel frattempo la Regione istituisce diciotto nuovi enti. Il disegno di legge, presentato inizialmente dal Consiglio regionale, prevedeva la modifica dello Statuto della Regione in materia di enti locali attraverso la sola soppressione delle Province. Nel corso del primo esame al Senato, con riferimento all'istituzione di nuovi Comuni, è stata prevista la possibilità che questi possano essere istituiti anche nella forma di Città metropolitane, con un'interpretazione, diciamo così, estensiva della volontà della stessa Regione, espressa all'unanimità, e allontanandosi dal modello della semplificazione, del risparmio e della sburocratizzazione. Questo mi induce ad una riflessione più generale sull'esorbitante numero di Città metropolitane partorite dalla riforma Delrio, che appare caotica e insoddisfacente per almeno tre motivi. In primo luogo, ha previsto l'automatica trasformazione di interi territori provinciali in Città metropolitane senza alcuna considerazione per criteri più oggettivi, quali i livelli di popolamento e urbanizzazione, attrazione di flussi di pendolarismo e di mobilità in generale, presenza di funzioni produttive di pregio. In secondo luogo, ha introdotto la possibilità di accrescere a dismisura il numero delle Città metropolitane. Infine, attribuisce di fatto al nuovo ente le stesse funzioni delle Province, con poche competenze aggiuntive e prevede un meccanismo di governo debole affidato a un Consiglio metropolitano formato da un sottogruppo di sindaci e consiglieri di tutti gli enti coinvolti. Viene così snaturato lo stesso concetto originario, sui cui si discute fin dal 1990, di Città metropolitana, che diventa un mero luogo di concertazione fra i Comuni, ognuno dei quali resta titolare delle proprie funzioni sul proprio territorio. Per una riforma il cui obiettivo è rilanciare la competitività del Paese attraverso il miglioramento dell'efficienza istituzionale il risultato è decisamente modesto. Più in generale, è tutta la riforma delle Province che sta facendo acqua, perché le Province non sono state abolite in attesa della riforma costituzionale: è stato di fatto moltiplicato il numero degli amministratori locali e sono stati determinati aggravi di costi, paralisi amministrativa e complicazioni decisionali. Non tutte le riforme, dunque, hanno di per sé implicazioni positive. Il disegno di legge costituzionale che abolisce le Province in Friuli-Venezia Giulia ha per lo meno il merito di abolirle davvero, anche se è prevedibile una fase di passaggio di consegne fra enti di complicata attuazione, che auspichiamo venga gestito meglio di quanto avvenuto a livello nazionale. L'abolizione delle Province va comunque nella direzione auspicata da quasi tutte le forze politiche e, quindi, tenuto soprattutto conto del fatto che il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia si è espresso all'unanimità su questo punto, annuncio il voto favorevole del Gruppo ALA.

vista degli assetti istituzionali e di governo del territorio che, credo, produrrà, a nostro avviso, molte difficoltà in futuro. Per tutti questi motivi, esprimeremo un voto di astensione.

il merito non è particolarmente interessante e questo è anche un motivo per essere rapidi. Si tratta semplicemente dell'adeguamento del regime autonomo del Friuli-Venezia Giulia ai principi della cosiddetta legge Delrio. Quello che è molto interessante, in realtà, su questa materia è il procedimento e tutto ciò che sta dietro a una modifica che, nel merito, non è poi affatto contestata. Nel merito si può forse semplicemente dire, molto brevemente, quanto sarebbe interessante e utile che una competenza quale quella che le Regioni a Statuto speciale hanno per l'ordinamento dei propri enti locali

A maggior ragione, quindi, sarebbe importante che anche le Regioni a statuto ordinario potessero dotarsi di questa competenza. Per fortuna, almeno le regioni a Statuto speciale ce l'hanno e non è appunto particolarmente contestato il fatto che ci si adegui ad un principio su cui c'è un vasto consenso. La questione di fondo riguarda il procedimento di revisione degli Statuti speciali.

data dalla necessità di avere una maggioranza costituzionale in Parlamento? Oppure questa maggioranza può comunque superare anche i limiti del principio pattizio, che sta pure alla base dell'autonomia speciale, il principio di sovranità del Parlamento? Forse alcuni ricorderanno ciò che è successo proprio con la proposta di modifica, strutturale in questo caso, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, elaborata anche con una convenzione regionale, poi fatta propria dal Consiglio regionale e infine presentata al Parlamento e poi assolutamente massacrata in Parlamento e arenatasi completamente. Questo era stato, tra l'altro,

neanche questo, grazie a queste rigidità procedurali. Ciò ha comportato, evidentemente, la creazione di un problema con le autonomie speciali in questo Paese. Tutti gli statuti ordinari sono stati modificati dopo la revisione del Titolo V nel 2001. Nessuno Statuto speciale è stato modificato. Questo ci dovrebbe fare un po' riflettere. Il problema si porrà soprattutto con la riforma costituzionale, se questa dovesse entrare in vigore. Pur prevedendo una clausola ancora più favorevole alle autonomie speciali, perché la revisione degli statuti avverrà previa intesa, si pone il problema se quest'ultima possa rappresentare un veto assoluto da parte delle autonomie speciali, oppure se il Parlamento debba comunque mantenere l'ultima parola Serve quindi una procedura unitaria per la revisione degli statuti o no? Come si garantisce l'equilibrio tra il principio pattizio, da una parte, che anche per giurisprudenza costituzionale e per dottrina unanime, sta alla base della specialità, con il specialità, con il principio di sovranità del Parlamento dall'altra parte? È difficile porre in capo ad un Consiglio regionale il potere di veto assoluto rispetto a modifiche votate con una maggioranza qualificata dal Parlamento medesimo. Evidentemente esiste una all'interno del nostro ordinamento che, in qualche modo, prima o poi dovrà essere affrontata. In questo caso, il problema non si pone. Questo testo è largamente condiviso nel merito, è anche compromissorio nella procedura, perché risulta dalla fusione di un testo di iniziativa del Consiglio regionale e di un testo di iniziativa però il problema che manca, e nella discussione sulla riforma costituzionale lo abbiamo visto in maniera molto grave, una concezione sistemica della specialità che pure riguarda il 20 per cento delle Regioni, il 15 per cento della popolazione quasi il 25 per cento della superficie del territorio nazionale. Questo tema è estremamente importante. Non è questa la sede per approfondirlo, ma almeno può essere un'utile occasione di richiamo ad una lacuna, anche concettuale, che ci stiamo portando dietro da troppo tempo e che sarebbe

motorizzazione civile, eccetera), alle quali ha fatto seguito un aumento delle risorse a loro disposizione. La cosiddetta legge Delrio ha ridefinito totalmente il ruolo delle Province, individuandole come enti di area vasta con funzioni fondamentali proprio legate alla programmazione e pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica, eccetera. Dunque, si tratta di enti sostanzialmente con un ruolo di servizio verso le comunità locali e i loro cittadini, da un lato, e verso i Comuni e gli altri enti locali, dall'altro. Il disegno di legge costituzionale in esame è volto a modificare lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia al fine di eliminare ogni riferimento al termine Provincia e realizzare un sistema di pubblici poteri locali fondato su due soli livelli di governo politico: la Regione e i Comuni. Il disegno di legge interviene, quindi, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. È da rilevare che il Friuli-Venezia Giulia ha la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Tale potestà esclusiva è vincolata unicamente all'osservanza di alcuni principi costituzionali e alle limitazioni cui soggiace anche il legislatore statale. Il testo del disegno di legge in oggetto è stato approvato dal Consiglio regionale nel gennaio 2014 con l'unanimità dei voti. Durante l'esame in prima lettura la Commissione ha svolto sulla materia un ciclo di audizioni informali, soprattutto in ragione dei molteplici profili riguardanti il rapporto tra fonti del diritto e, più in particolare, il peculiare procedimento previsto per le modificazioni degli Statuti speciali. All'esito di questa fase istruttoria e a conclusione della discussione generale, si è deciso di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge costituzionale n. 1289, di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Con tale intervento normativo si intende realizzare un sistema istituzionale dei pubblici poteri locali più razionale, fondato su due livelli di governo politico, espressione della sovranità popolare: la Regione e i Comuni. L'approvazione parlamentare di tale riforma permetterà di procedere ad un incisivo cambiamento dell'assetto istituzionale, in cui i livelli essenziali dei servizi resi alla comunità possano essere meglio garantiti da aggregazioni territoriali in grado di contemperare il principio di sussidiarietà con quelli della differenziazione, costituzionalmente sanciti, e di armonizzare le ragioni dell'autonomia locale con quelle della semplificazione e dell'efficienza. Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Gruppo Area Popolare voterà a favore del provvedimento. Presidente, abbiamo una buona notizia, perché il sottosegretario Bressa finalmente ammette la bugia del Governo: le Province non sono abolite, ma trasformate.

manterrà il 90 per cento dei suoi costi e sarà semplicemente sottratto alla volontà dei cittadini elettori.

non dice che l'*iter* di questo disegno di legge ha visto ledere la volontà popolare espressa dai rappresentanti dei cittadini friulani e giuliani, che hanno proposto al Parlamento un disegno di legge. Ma questo Parlamento e questa maggioranza si sono sentiti in dovere di peggiorare quel testo. L'esame legislativo, infatti, si è attivato a seguito di una proposta di legge d'iniziativa della stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base di un documento che quella stessa assemblea aveva votato unanimemente, dal PD al Movimento 5 Stelle, da SEL a Forza Italia, passando per le altre liste civiche. In quella proposta di legge si procedeva a riconoscere solo due livelli amministrativi e di governo territoriale: la Regione e il Comune. Invece avete voluto inserire un nuovo terzo livello: la Città metropolitana; anzi, le Città metropolitane, perché il testo apre alla possibilità indeterminata di avviarne anche delle altre. una Città metropolitana voluta solo dal Comune di Trieste, che sarà egemone e disomogeneo rispetto agli altri piccoli Comuni inglobati, che vogliono mantenere la propria autonomia ed indipendenza territoriale e politica nella gestione del territorio, perché hanno una realtà urbanistica diversa, una dimensione diversa anche dal punto di vista culturale, perché in questi Comuni vige il bilinguismo.

carta canta e villan dorme! Peraltro, abbiamo già visto (e ne abbiamo una conferma) l'attitudine del Partito Democratico a nominarsi da solo i rappresentanti nelle istituzioni, dimostrando di voler ridurre sempre più la volontà popolare. Anche la riforma costituzionale, infatti, bocciata da quasi tutti i maggiori costituzionalisti italiani (ex presidenti della Corte costituzionale, magistrati, professori universitari dei maggiori atenei del nostro Paese) prevede, come sappiamo, un Senato nominato dai Consigli regionali. La riforma delle Province e delle Città metropolitane ha previsto che i relativi consigli siano nominati dagli stessi consiglieri comunali già eletti nelle Province (eletti che nominano eletti). Tuttavia, in questo passaggio i giochi di potere delle segreterie avranno controllo su tutto, dunque in sfregio ai principi della Carta europea dell'autonomia locale, sottoscritta dall'Italia nel 1985 e ratificata con la legge n. del 1989 che, all'articolo 3, stabilisce che i consigli e le assemblee delle autonomie locali siano costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale. La seconda conferma riguarda l'atteggiamento schizofrenico del Partito Democratico, spaccato al suo interno e frantumato tra livello nazionale e territori, come dimostra da ultimo l'esperienza del *referendum* sulle trivellazioni petrolifere, voluto da molte Regioni a maggioranza PD e osteggiato dalla segreteria nazionale del PD stesso. Analogamente, in Friuli-Venezia Giulia, Regione governata dal suo vice segretario nazionale nonché esponente di punta di quel partito, Debora Serracchiani, il PD vota un testo e il partito nazionale lo stravolge. caso siamo proprio al paradosso perché, dopo le modifiche, il Consiglio di una Regione a statuto autonomo non è stato nemmeno degnato di un passaggio istituzionale. 5 Stelle la linea è chiara: ci siamo sempre opposti e continueremo a farlo, non solo in Friuli-Venezia Giulia, agli organi istituzionali intermedi tra Comuni e Regioni e riteniamo che siano sempre i cittadini a dover eleggere i propri organi legislativi e amministrativi. metropolitana (delle Città metropolitane), si va ad aggiungere un'altra beffa, di cui accennavo, introdotta con legge regionale, quella delle UTI (Unioni territoriali intercomunali), che non sono le unioni tra Comuni, ma enti stabiliti dalla Regione, definiti dall'alto, come dall'alto viene stabilita la figura del direttore generale, una persona la cui retribuzione raggiunge i 150.000 euro l'anno. Era utile fare chiarezza, escludere esplicitamente la reintroduzione delle Province camuffate e di questi altri enti intermedi, come le UTI, e, invece, signor Presidente, su questo disegno di legge sono state apportate modifiche opposte. Queste modifiche, così come il metodo centralista utilizzato per apportarle, non possono non incidere sul giudizio di un testo che, in origine, aveva anche delle innovazioni apprezzabili; mi riferisco all'abbassamento da venticinque a diciotto anni del limite di età per poter essere eletti

queste che potevano risultare migliorie appaiono, purtroppo, come compensazioni troppo parziali. In ragione di ciò, il Movimento 5 Stelle dichiara dunque il suo voto di astensione.

abolisce, così almeno dice il titolo (ma come spesso accade per le leggi di questo Governo, il titolo contiene qualcosa di allettante, poi il testo è ben diverso) - le Province. Ma se dovesse - per disgrazia generale e non certo per il problema delle Province *-* essereapprovato il *referendum* costituzionale,

In secondo luogo, abbiamo - e anche questo è interessante per tutta l'Italia, non certo solo per il Friuli-Venezia Giulia - un assaggio di quello che accadrebbe se passasse questo tipo di riforma dell'ordinamento degli enti locali

18 Unioni territoriali intercomunali, che non si chiamano effettivamente più Province, ma sono la stessa cosa. Attualmente, in tutta l'Italia, c'è solo un ente

mediamente governerà poco più di 60.000 abitanti (perché questo avverrà) e probabilmente anche meno, perché mi sembra difficile che si voglia frazionare la città di Trieste,

Ma non bastano le "unionine territorialine intercomunaline"; ci sarà anche la Città metropolitana, che è stata rifiutata in Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, ma che viene introdotta in Pare di capire che sia destinata a Trieste, città di grande prestigio, importantissima nella nostra storia, però di 200.000 abitanti. Nel resto d'Europa, che io sappia, ci sono nove o dieci

che è capoluogo di una delle quattro "abolende" Province, ha la bellezza di 35.000 abitanti; si potrebbe fare una bella Città metropolitana di 35.000 abitanti: Londra, Parigi e Gorizia (lo dico sempre con grande rispetto per questa importante città che è cara a tutti noi italiani).

la Città metropolitana ipotizzata per Trieste non avrebbe l'assurda e mostruosa conformazione che hanno le Città metropolitane volute dalla legge

per cui c'è un sindaco metropolitano (già il nome è abbastanza strano), che può essere sfiduciato non dalla Città metropolitana ma solo dal Consiglio comunale. Infatti abbiamo sostanzialmente una metropoli

perché sarà necessaria la doppia maggioranza per cui ci sarà il rischio che i pochissimi altri Comuni che non sono Trieste potranno imporre la propria volontà al Comune di Trieste. Si tratta di un pasticcio straordinario al quale Forza Italia dirà "no"

queste 18 Unità territoriali intercomunali vengono imposte ai Comuni. Alcuni Comuni si sono rifiutati di entrare in questi agglomerati forzosi

e tagli dei trasferimenti. Direi che si tratta di una procedura inaccettabile e di un risultato risibile e probabilmente peggiorativo che si aggiunge al pasticcio della legge nazionale che ha malamente riformato le Province. Comunque, ribadisco, questo testo ha un pregio: ci dice come funzionerà la cosiddetta abolizione delle Province a livello nazionale: avverrà la loro moltiplicazione per quattro. A tutto questo noi diciamo no. *(PD)*. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della riforma dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia lo farà convinto dell'importanza che le autonomie speciali hanno nel riordino del nostro sistema autonomistico.

In particolare, le autonomie speciali del Nord sono servite a gestire in modo brillante due questioni molto complesse. La prima è quella della convivenza tra popolazioni di lingua diversa, in zone di frontiera che hanno lacerato l'Europa nel secolo che abbiamo alle spalle.

tedesca-austriaca-mitteleuropea e quella slava. Si tratta di luoghi che sono stati teatro di tragedie immani nel secolo che abbiamo alle spalle: la Prima guerra mondiale e poi la Seconda guerra mondiale, con tutti gli strascichi che conosciamo le autonomie speciali hanno saputo gestire brillantemente tali questioni e sono diventate un vanto per il nostro Paese: la via italiana alla soluzione di questi problemi. L'altra grande questione che hanno saputo affrontare è stata quella delle genti di montagna. Hanno saputo cioè gestire il passaggio da una fase nella quale montagna voleva dire sottosviluppo ad una fase nella quale montagna può voler dire un modo diverso Nel caso del Friuli, abbiamo poi questo abbinamento tra la montagna e il mare, il porto, l'apertura nell'Adriatico. Ebbene, rispetto a tali questioni siamo in una fase di discussione approfondita sul futuro delle nostre istituzioni. Siamo ormai nel pieno di un confronto referendario sul futuro della nostra Costituzione e gli Statuti speciali fanno parte di questo patrimonio costituzionale del nostro Paese; essi sono quindi parte della nostra discussione. Io penso che il voto di oggi voglia dire che noi continuiamo a credere nelle autonomie speciali, ad alcune condizioni naturalmente. La più importante è che le autonomie speciali si vivano come un laboratorio di sperimentazione di soluzioni più avanzate e non come un luogo di freno e di chiusura rispetto al cambiamento. La seconda è che facciano proprio l'ammonimento di Alcide De Gasperi, nella discussione in seno all'Assemblea costituente nel gennaio del 1948, quando il grande statista (fondatore, insieme ad altri, della nostra Repubblica) ammoniva le autonomie speciali a fondare la loro autonomia sulla capacità di fare meglio dello Stato, spendendo meno e costando meno dello Stato. Questo è un obiettivo che deve essere sentito come proprio da tutte le autonomie speciali.

il nuovo articolo 116 della Costituzione, come riformato dal Parlamento (adesso attendiamo il parere definitivo del popolo), del popolo), lascia immaginare, cioè un mondo di Regioni che collaborano con lo Stato nel nuovo Senato. Quest'Aula diventerà il luogo dell'incontro e del confronto tra il legislatore regionale e il legislatore statale, mentre nei diversi territori si sperimenteranno anche forme diverse di autonomia. Quindi il rapporto tra le autonomie speciali e le autonomie ordinarie cambierà, perché non ci sarà più quello scalino che oggi differenzia in maniera così netta una parte delle nostre autonomie dalle altre, ma ci sarà un *continuum*, dentro il quale diverse Regioni, ciascuna a modo suo, troveranno il loro spazio nel confronto tra loro e nel confronto con il Governo centrale. Ecco, è dentro questo percorso che si inserisce la riforma dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia che votiamo oggi, che ha al centro proprio il ridisegno del sistema dei poteri locali su due perni fondamentali, quello della Regione e quello dei Comuni. Si tratta quindi di un modello di semplificazione e di ammodernamento; è una direzione che va bene e che è in sintonia con l'orientamento generale del nostro Paese. Nutriamo questi sentimenti, questa speranza e questa fiducia nei confronti di questa importante Regione, che ha segnato pezzi decisivi della storia del nostro Paese, dalla Prima guerra mondiale ad oggi. Prima è stato ricordato giustamente il terremoto del Friuli. Resta ancora un *unicum* la capacità che ebbero quel popolo e la sua amministrazione autonoma di affrontare, con efficienza e umanità, quel passaggio così difficile. Siamo attenti osservatori di questo laboratorio importante e interessante per il nostro Paese, collocato in una zona di frontiera così decisiva, ed è per questo che voteremo a favore della proposta di modifica dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'articolo 138, primo comma della Costituzione, dovendosi procedere alla votazione di un disegno di legge costituzionale, in sede di seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta

Signor Presidente, senatrici, senatori, signor Sottosegretario, il disegno di legge in esame mira al rafforzamento delle politiche ambientali, consolidando e completando il percorso riformatore avviato con la legge n. 61 del 1994, grazie alla quale fu istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e vennero poste le basi per la costruzione di strutture, di competenze professionali e tecnologiche acquisite attraverso lo studio, l'analisi, il monitoraggio e il controllo dei dati ambientali. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in esame il 17 aprile 2014, in esito ad un'approfondita attività istruttoria, che ha consentito l'acquisizione di significativi elementi conoscitivi, anche grazie al contributo di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione. Il lavoro istruttorio svolto nelle audizioni ha rappresentato una risorsa per l'arricchimento del testo, con il contributo di riflessioni e di proposte, portate nel corso delle audizioni dai rappresentanti di AssoArpa, dell'Istituto dai rappresentanti di Legambiente, di Greenpeace, del WWF, dell'Associazione medici per l'ambiente, del Capo della Protezione civile, dei rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'ENEA e di Rete Imprese Italia. In questi due anni, dall'approvazione alla Camera dei deputati ad oggi, in materia ambientale sono successe molte cose e ne voglio ricordare in particolare due. La prima è la Conferenza internazionale sul clima di Parigi del dicembre del con l'approvazione dell'accordo internazionale sul clima, sottoscritto da quasi duecento Governi, tra cui quelli di Cina e Stati Uniti, i principali responsabili delle emissioni di gas serra. un accordo che entrerà in vigore nel 2020, con l'impegno dei Paesi firmatari a limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Sappiamo che non è sufficiente e che è necessario un maggiore impegno dei singoli Stati. Di sicuro, però, la Conferenza ha sollecitato e valorizzato l'attenzione dei cittadini sullo stato di salute dell'ambiente, sulle scelte alimentari, sullo sviluppo sostenibile, sull'agricoltura e sulla riduzione del consumo del suolo. secondo punto, nei mesi scorsi abbiamo approvato due leggi importanti ed attese, quella sui reati ambientali e il collegato ambientale. Ad entrambe questo provvedimento è strettamente legato: con la legge 22 maggio 2015, n. 68, si è introdotto nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai «Delitti contro l'ambiente» prevedendo nuove fattispecie quali l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico ed abbandono di materiale radioattivo, l'impedimento di controllo e l'omessa bonifica. Abbiamo riconosciuto all'ambiente il diritto di essere tutelato e quindi di punire più severamente questi reati. Coerentemente dobbiamo adesso attivare e garantire migliori controlli, più coordinati, puntuali ed efficaci, ed è questo l'obiettivo di questo disegno Con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015, il cosiddetto collegato ambientale, si sono introdotte norme sui rifiuti, bonifiche e rischio idrogeologico. Ai cittadini e alle imprese dobbiamo garantire che i controlli e le autorizzazioni su queste materie non vedano velocità e interpretazioni diverse nelle diverse aree del nostro Paese. Il disegno di legge si prefigge l'obiettivo del riconoscimento normativo del Sistema nazionale delle Agenzie per la protezione dell'ambiente e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento finalizzate - secondo quanto prevede l'articolo 1 ad assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. L'articolo 2 reca definizioni funzionali all'applicazione della legge, tra le quali in particolare la definizione di Sistema nazionale delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) disciplinati dall'articolo 9. Il quadro delle funzioni di indirizzo e coordinamento prevede l'elaborazione di criteri e *standard* uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo della prevenzione rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico. L'articolo 5 prevede di trasferire all'ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino. Tali funzioni sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della legge. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4, i componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Identica durata è prevista

Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono stati specificati, all'articolo 8, i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle Agenzie per la protezione Inoltre, è previsto che presso l'ISPRA sia istituita e costantemente aggiornata un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali e provinciali, che contiene le informazioni sui requisiti professionali e sullo stato patrimoniale dei direttori delle medesime Agenzie. L'articolo 7, comma 1, attribuisce anche alle Agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le leggi regionali disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle Agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'articolo 10. L'articolo 9 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. Al riguardo, è opportuno richiamare la definizione recata dall'articolo 2, comma secondo cui per livello essenziale di prestazioni e si intende lo *standard* qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambientale. Il comma 2 dell'articolo 9 infatti chiarisce che i LEPTA fissano gli *standard* funzionali, operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione del catalogo nazionale dei servizi: stabilire che esistano livelli essenziali di prestazioni tecnico-ambientali rappresenta la possibilità di omogeneizzare gli interventi in tutte le Regioni, garantendo a tutti i cittadini lo stesso livello e la stessa qualità di prestazioni in campo ambientale. Sono inoltre disciplinate le modalità di aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, e comunque con cadenza non superiore a cinque anni. L'articolo 10 prevede una specifica programmazione triennale delle attività, mentre l'articolo 11 disciplina la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale. L'articolo 12 disciplina la rete nazionale dei lavoratori accreditati, mentre l''articolo 13 istituisce il consiglio del Sistema nazionale - presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA con funzioni consultive e parere vincolante su tutti gli atti di indirizzo e coordinamento per il governo del sistema, ivi compreso il programma triennale, nonché sui provvedimenti del Governo di carattere tecnico in materia ambientale e di segnalazione al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge. L'articolo 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema, favorendo il principio di rotazione del medesimo personale, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. L'individuazione del personale ispettivo è basata su principi di merito, e con il regolamento sono disciplinate le modalità con cui i cittadini segnalano presunti illeciti ambientali. I commi 5 e 6 disciplinano i poteri del personale ispettivo, mentre il comma 7 dispone che il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie possono individuare, nell'ambito del personale incaricato degli interventi ispettivi, quelli che operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Inoltre, l'articolo 17 reca una disposizione che è stato necessario inserire in sede referente, a seguito del parere della Commissione bilancio, che ha subordinato l'espressione dell'avviso favorevole a condizione che il disegno di legge recasse una clausola complessiva di invarianza finanziaria.

Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati a discutere, in prima lettura, del disegno di legge in materia di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, La Commissione ambiente del Senato ha approvato una modifica concernente l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria: l'unico e significativo ritocco, vista la pochezza di ulteriori variazioni apportate a una tematica già rispolverata più volte. Questa clausola è stata apposta per permettere il recepimento, in base all'articolo 81 della Costituzione, di una condizione posta dalla Commissione bilancio del Senato; una scelta inaccettabile, a mio avviso, poiché si vuole concepire una nuova riformulazione delle Agenzie percorrendo l'istituzione di un Sistema nazionale a rete senza stanziare le risorse vitali a tal fine. Nel dettaglio, il disegno di legge riguarda, appunto, l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente; inoltre, disciplinerà l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, meglio conosciuto con l'acronimo di ISPRA. Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente è composto anche dalle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. L'istituzione del Sistema nazionale mira al riconoscimento normativo del tratto distintivo sistematico delle Agenzie ambientali, e all'ingresso di concrete innovazioni organizzative e di funzionamento che mirino ad assicurare omogeneità ed efficacia allo svolgimento dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente. Tutto questo va a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. L'istituzione dell'ISPRA, come concepita dalle modifiche del disegno di legge al nostro esame, è la raffigurazione di una struttura centralista che non contempla minimamente le diversità ambientali che si possono riscontrare a livello regionale. L'ISPRA e l'eventuale Sistema nazionale a rete non tengono conto delle ineguali esigenze territoriali di ogni singola Regione, ed è ingiustificabile che tutto ciò possa essere riportato su scala nazionale in maniera omogenea per quanto concerne le attività qualitative e quantitative. Il testo in esame contiene al suo interno molte novità. In primo luogo, vengono istituiti i LEPTA. Molti di voi, colleghi, si domanderanno che cosa sono: non sono altro che livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali garantiti dal Sistema nazionale, che andranno a creare un termine di raffronto imprescindibile per la pianificazione delle attività delle Agenzie. Il Sistema sarà integrato con diversi compiti, che si trovano racchiusi all'interno dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, i quali possono essere riassunti in: monitoraggio dello stato dell'ambiente; controllo dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. L'articolo 4 disciplina le funzioni dell'ISPRA e i profili di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. L'ISPRA riceverà anche le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente per i quali era stato avviato un procedimento di riordino. Mi soffermo, in ultimo, sulle Agenzie per la protezione dell'ambiente, la cui struttura interna e i cui compiti saranno di competenza regionale.

dell'ambiente avranno libertà di svolgere ulteriori attività, con la limitazione di non interferire con il raggiungimento finale dei LEPTA. Se esse svolgeranno attività per soggetti pubblici o privati, suddette attività dovranno essere compatibili con l'obbligo di imparzialità nell'esercizio delle attività di vigilanza e di controllo. Concludo, esprimendo forti dubbi sulle modalità e le valutazioni di alcuni punti del presente disegno di legge. Positiva è solo l'intenzione di creare un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ma scritta e realizzata male. Auspichiamo che attraverso la disciplina degli strumenti di partecipazione pubblica si possa raggiungere un'uniformità tra le parti,

solidarietà, come Sinistra italiana, ai lavoratori e ai ricercatori dell'ISPRA, che in questo momento sono a difendere - anche questa mattina erano sotto il Ministero dell'ambiente

d'istituzione del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente, che riconosce all'ISPRA un ruolo fondamentale di coordinamento delle ARPA per garantire al Paese un'omogeneità di

Non vorremmo parlare di bancarotta, ma siamo molto preoccupati. Tra l'altro, le prime vittime di questa situazione rischiano di essere quei ricercatori precari che lavorano ormai da anni e che hanno fatto la storia anche scientifica dell'ISPRA, che hanno lavorato per i *report* annuali, che, per esempio, ci hanno detto della contaminazione di pesticidi - è notizia di questi giorni - nelle acque

alla discussione dell'Aula, ma, a nostro avviso, è sostanzialmente positivo e riforma finalmente il settore delle Agenzie ambientali, sia quelle regionali che nazionali, istituendo il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, cui vengono affidate funzioni di indirizzo, coordinamento tecnico, controllo, monitoraggio, ricerca, consulenza tecnica e formazione e disciplinando l'ISPRA. Per questo penso che dovremmo rivolgere una particolare attenzione a quello che sta accadendo. La prima legge in materia - vorrei ricordarlo - è di più di venti anni fa e istituì l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali, a seguito di un *referendum* che tolse ai presidi

Purtroppo, gli enti locali e le Regioni si sono tutti adeguati con estrema lentezza. Tutto questo in questi venti anni è stato costellato, nella storia del nostro Paese, da drammatiche e continue vicende legate ai disastri ambientali, che via via hanno messo in evidenza le resistenze nei confronti di un pieno sviluppo dei sistemi di analisi, monitoraggio e controllo ambientali. Tutto questo è accaduto, per fortuna, in un contesto di crescente consapevolezza e richiesta da parte dei cittadini di un reale accesso alle informazioni ambientali, riconosciuto - lo vorrei ricordare - a livello internazionale e comunitario come diritto inscindibile dal diritto all'ambiente e alla salute. Ricordo, oltre alla Convenzione come la Francia abbia inserito in Costituzione tale diritto già nel 2004 attraverso la Charte de l'environnement. Sottolineo, inoltre, come l'accesso ai dati e alle informazioni ambientali è assolutamente complementare al diritto di partecipare ai processi decisionali che impattano sull'ambiente. L'elemento dell'informazione, dell'accesso dei cittadini all'informazione e della partecipazione è assolutamente inscindibile dal diritto all'ambiente. È evidente che, in tale contesto, era ed è ancora di più oggi necessario garantire l'autorevolezza delle informazioni che vengono acquisite e divulgate ai cittadini, anche per assicurare una piena comprensione del legame esistente tra i valori ambientali ed i fattori di rischio per la salute. Una delle maggiori criticità manifestatasi negli anni è stata proprio la profonda disomogeneità tra funzioni, risorse e meccanismi delle varie Agenzie regionali. Basti pensare che al Nord, il personale addetto al monitoraggio ambientale controlla 131 chilometri quadrati di territorio, mentre al sud 345. È evidente, dunque, come una riforma in questo senso sia assolutamente necessaria. È quindi positivo che in questo provvedimento vengano individuati i livelli essenziali di prestazioni in materia di ambiente (i LEPTA), ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, quale livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, e che tali livelli debbano essere attuati dal Sistema nazionale nel suo insieme (ISPRA e Agenzie regionali). L'ISPRA predisporrà un programma triennale delle attività del Sistema nazionale, individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.

Tra l'altro, nonostante già nel provvedimento approvato dalla Camera fosse chiaro che c'era una clausola di invarianza finanziaria, si è voluto di nuovo ulteriormente ribadirlo anche nel passaggio al Senato,

Peraltro, nessun altro emendamento è stato approvato in Commissione. Le opposizioni si sono fatte carico anche di fare in modo che ci fosse effettivamente un'approvazione; ci troviamo invece di fronte di una parte del Governo non certamente favorevole al provvedimento. Come si può pensare di procedere alla riorganizzazione e al rafforzamento di un sistema tanto complesso e necessario senza la previsione di nuove risorse? L'articolo 15, relativo alle modalità di finanziamento, prevede infatti che l'ISPRA e le Agenzie provvedano alle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questo è un punto, e lo dico alla relatrice, che noi, magari anche con un impegno rispetto alla prossima legge di stabilità, dobbiamo assolutamente affrontare. Così come dobbiamo affrontare la situazione grave, dal punto di vista finanziario, dell'ISPRA.

infatti quasi inutile quanto previsto dall'articolo 16, ove si dispone che l'ISPRA e le Agenzie possano procedere all'assunzione di personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali.

in materia di assunzione relativi al Patto di stabilità a non consentire la stabilizzazione del personale che conduce quotidianamente un compito così delicato. Nuovamente, dunque, penso che al Governo manchino il coraggio e la volontà per rendere pienamente soddisfacenti e operativi provvedimenti che vengono sentiti come un'esigenza forte da parte della società. Pertanto, spero che nell'esame ulteriore del provvedimento il Governo metterà in campo

la necessità di un riordino del sistema delle Agenzie ambientali è determinata sia dalla datazione della normativa vigente, risalente al 1994, sia dalle sopravvenute normative comunitarie e nazionali, che hanno profondamente modificato il diritto ambientale e riformato la pubblica amministrazione. Il gruppo Lega Nord e Autonomie condivide l'obiettivo primario del provvedimento in esame, che è quello di garantire un'articolata ed omogenea disciplina per le attività delle ARPA e porre fine alla situazione attualmente esistente nelle diverse aree del Paese, anche sul piano normativo, che vede alcune ARPA svolgere controlli serrati e applicare norme rigide agli operatori e agli impianti e altre Agenzie addirittura chiudere gli occhi davanti a evidenti situazioni imbarazzanti, illegittime e dannose per l'ambiente e, soprattutto, per la salute dei cittadini. Penso, solo per citare qualche esempio, alla cosiddetta terra dei fuochi in Campania, all'inquinamento ambientale dell'ILVA di Taranto, proseguito nell'indifferenza per anni, e allo scandalo petroli in Basilicata. è avvenuto perché ciascuna Regione ha provveduto a istituire la propria Agenzia nella massima autonomia e in modo differenziato e, quindi,

Concordiamo, dunque, sul fatto che esistono aspetti del sistema delle Agenzie che occorre riorganizzare e razionalizzare e che occorre finalmente stabilizzare molti aspetti lasciati eccessivamente sospesi dal 1994.

e secondo i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). Ciò - si spera - dovrebbe garantire alti livelli di qualità ambientale a tutti i cittadini, evitando così anche una concorrenza sleale tra gli operatori, in considerazione degli alti costi ambientali richiesti per la messa a norma degli impianti. Entrando nel merito del provvedimento in esame, il disegno di legge approvato in prima lettura alla Camera dei quindi oltre due anni fa, peraltro con un'ampia convergenza, ha certamente molti aspetti innovativi e condivisibili.

A nostro avviso, doveva essere intrapreso un esame sereno delle lacune del testo alla luce delle moltissime criticità della realtà ambientale in cui viviamo e di quelle oggi presenti nelle Agenzie ambientali e, soprattutto, realtà che, giorno dopo giorno, in tutte le Regioni, soprattutto del Centro-Sud, emergono mettendo a nudo situazioni critiche, preoccupanti e talvolta allarmanti in tema ambientale, con conseguente riflesso sulla salute. A queste criticità del testo doveva necessariamente corrispondere l'accoglimento di proposte emendative, peraltro considerate apprezzabili sia dal relatore che dal Governo in Commissione, molte delle quali avanzate dal Gruppo della Lega Nord. Ancorché non sussisteva motivo in ordine alla necessità di licenziare velocemente il provvedimento blindato per evitarne il ritorno alla Camera, visto che il testo

finale di invarianza finanziaria introdotta, deve ritornare necessariamente a Montecitorio. Si doveva - e auspico si possa ancora cogliere l'opportunità connessa alla schizofrenia - e ripeto schizofrenia - della Ragioneria generale dello Stato, che un anno fa dava indicazione di mettere la clausola di invarianza finanziaria in diversi articoli del provvedimento e ora invece si sveglia prevedendone una finale e complessiva, creando un testo pasticciato, zeppo di clausole di invarianza finanziaria tanto nei vari articoli quanto nella parte finale del testo.

È stata imboccata la strada della definizione di meccanismi trasparenti e oggettivi per il finanziamento delle Agenzie, ma in pratica si è rinunciato a garantire i finanziamenti per un periodo indefinito. Sul punto deve essere chiaro a tutti che da questa rinuncia consegue in automatico la rinuncia alla verifica della corretta erogazione da parte delle Agenzie del compito che i cittadini da esse si aspettano, soprattutto dopo le tante tasse versate. Non investire nel settore e non considerare la qualità ambientale come un valore capitale per il progresso e il benessere anche economico dell'Italia non solo è un atteggiamento poco lungimirante, ma di fatto tutela altri interessi, con evidenza di *lobby* e di quanto c'è di più illecito, pericoloso e dannoso in Italia, come deriva anche dalla mia esperienza di componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti. Mi domando, però, come saranno garantiti i controlli obbligatori

evidenzia è legato al carattere centralista del provvedimento, visto il ruolo centrale che si vuole affidare a ISPRA rispetto alle Agenzie territoriali. Questo è certificato dalla previsione del ruolo organizzativo di ISPRA sulla definizione delle attività che si svolgono sul territorio e l'attribuzione del ruolo di coordinamento centralizzato della programmazione delle Agenzie regionali in ordine all'attività di monitoraggio, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale. L'approccio omogeneo alla protezione dell'ambiente in tutte le realtà territoriali è condivisibile. Ma, alla luce dell'esperienza quotidiana, deve trovare un riscontro molto più adeguato, realistico ed efficace, che tenga conto delle maggiori competenze tecniche e operative acquisite sul campo dalle varie Agenzie; competenze e *know-how* che, con il nuovo testo, rischiano di perdersi. Sottolineo la riforma, non mettendo mano alla struttura di ISPRA, non può essere un mezzo per farle riguadagnare, in forza di legge, il ruolo che non è stata in grado di svolgere in tutti gli anni di esistenza dal 1994, anno della sua prima istituzione, Peraltro, un altro aspetto critico che riguarda l'ISPRA è il mantenimento della natura di istituto di ricerca. La nuova legge non interviene sui compiti di ricerca dell'Istituto e senz'altro l'accavallamento delle competenze aggraverà ancora di più i problemi impattanti sulla struttura organizzativa in termini di razionalizzazione ed efficienza e le proteste in corso dei ricercatori lo stanno a dimostrare. La terza e ultima criticità che voglio rilevare in discussione generale e che generale e che la proposta di legge non risolve è il tema del rapporto tra Agenzie e imprese. Il tema della promozione della qualità ambientale, elemento essenziale anche nelle politiche europee nel quadro della gestione delle pressioni ambientali, è trattato marginalmente e poco concretamente. È evidente che il tema del rapporto tra ambiente e salute implica conseguentemente il rapporto delle Agenzie per la con il Servizio sanitario. Qui dobbiamo auspicare la migliore integrazione delle attività di queste strutture e, dove utile e ne ricorrano le condizioni, l'ottimizzazione delle risorse a disposizione. avvenire nella massima chiarezza dei ruoli e nel chiaro privilegio, per le Agenzie, della missione affidata loro dalla legge n. 61 del 1994. Non si tratta di erigere barriere o spaccare il sistema della prevenzione, ma semplicemente di esplicitare quali sono i compiti di competenza propri delle strutture sanitarie che che trovano spesso attuazione solo attraverso un impegno delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, con ciò sottraendo risorse alle loro funzioni primarie. Si tratta, insomma, di operare perché i compiti delle strutture sanitarie siano effettivamente e completamente assolti, anche nel campo della prevenzione, come dalle aspettative dei cittadini e dal dettato della Costituzione, senza che le Agenzie per la protezione dell'ambiente siano chiamate a metterci ancora una volta una pezza. Mi avvio alla conclusione dicendo che, scontata la blindatura del testo, auspichiamo, come Gruppo Lega Nord-Autonomie, che almeno la maggioranza e il Governo possano accogliere gli ordini del giorno presentati dal nostro Gruppo, perché da ciò dipenderà il nostro voto finale sul provvedimento. *(Applausi

Sono profondamente convinto che la tutela dell'ambiente sia una delle priorità per ogni persona che vive su questa terra; una terra che ci è stata donata da Dio e che sarebbe nostro dovere primario difendere in suo nome, dal momento che la relazione con il creato è elemento fondamentale dell'identità umana stessa, come frutto del rapporto, ancor più profondo, dell'uomo con Dio. Lo stesso Gesù ci ha donato parabole in cui la natura faceva da cornice mirabile e poetica, ma anche da necessario complemento alle giuste azioni di un uomo che cerca la verità in Dio. Come si legge nel Vangelo secondo Marco, nel suggestivo passaggio della tempesta sedata, chi è pieno di Spirito Santo è anche il grado di ammansire la natura, creando un rapporto di convivenza fatto di amore e rispetto reciproco, perché il Padre ci ha donato un giardino affinché sia coltivato e custodito, così da preparare la venuta del suo regno di pace in cui il suo popolo vivrà in eterno. Ma ciò che mi spinge da sempre all'assoluta attenzione ai problemi ambientali non è certo solo la mia fede cattolica e cristiana. Ritengo ancora che si debba decisamente invertire la tendenza, mantenendo con forza il nostro Parlamento e il Governo laico, focalizzando l'attenzione su quei principi e valori cristiani da difendere strenuamente e senza titubanza. È anche la certezza che il territorio debba essere difeso, sempre e comunque, perché si tratta di una vera e propria ricchezza, nonché nostra dimora terrena, ed è l'unica possibilità che esista per tutelare la vita stessa. Questo è vero a maggior ragione per il nostro Paese, in virtù delle sue bellezze naturali, storiche e artistiche e della tradizione culturale che rappresenta nel mondo. L'assalto ambientale che vediamo quotidianamente attraverso l'inquinamento, la proliferazione inconsulta del cemento e il mancato rispetto delle leggi esistenti è un attentato non solo al nostro futuro, ma anche alla nostra ricchezza. L'Italia deve avere ben chiaro che, in un mondo occidentale che vive ormai da anni una crisi sistemica e - ho paura persino a dirlo - irreversibile, la grandiosità e la varietà del nostro territorio possono essere un elemento cardine, se ben sfruttato, per lo sviluppo futuro del nostro Paese. È partendo da questo punto di vista che si deve valutare il disegno di legge Come tutti voi sapete, questo provvedimento ha due cardini fondamentali: l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e una nuova disciplina per l'ISPRA, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale. Sulla prima questione, vorrei innanzi tutto ricordare che il Sistema nazionale delle Agenzie ambientali è stato accorpato, per la prima volta, proprio dal Governo Berlusconi nel 2008. In questo nuovo assetto, il Sistema nazionale acquisisce una serie di funzioni molto importanti, tra cui concorrere a uno sviluppo sostenibile e alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, alla riduzione del consumo del suolo e alla realizzazione piena e completa del principio che chi inquina paga. In più, nuocere consapevolmente a un proprio fratello è colpa ancora più grave perché Gesù ha detto: «ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me», nel bene e soprattutto nel male. La vita è sacra perché anche in quella che apparentemente risulta più insignificante vi è sempre la presenza di Cristo, in quanto siamo tutti fratelli e figli dello stesso Dio. Nel nuovo assetto ha inoltre una importantissima funzione l'articolo 2. Sta, infatti, alla rete il compito di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, cioè quel livello minimo di una serie di attività come il monitoraggio ambientale, il controllo delle fonti di inquinamento, le attività di ricerca e tante altre cose che vengono indicate nell'articolo 3 e devono essere omogenee su tutto il territorio nazionale. Ricordo che, a tal proposito, avevo presentato una proposta di legge, la n. 368, intitolata: «Delega al Governo per l'adozione di norme a salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento nelle zone interessate da impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani ed industriali», nel lontano 5 giugno 2013. Tale proposta, purtroppo, risulta ancora inascoltata. La rete per la protezione dell'ambiente, quindi, viene indicata come l'autorità che avrà il compito di coordinare le attività di tutte le Agenzie ambientali, ma anche come primo motore per un efficace sistema di controllo e di monitoraggio del territorio italiano. La seconda parte del provvedimento - come abbiamo già detto - riguarda l'ISPRA, definendone una nuova personalità giuridica, ossia società di diritto pubblico, disciplinandone l'autonomia tecnico-scientifica e specificando i suoi profili di ricerca, organizzazione e autonomia patrimoniale e contabile. Ma il disegno di legge non si limita agli aspetti organizzativi e societari. Esso affida, infatti, all'Istituto superiore per la protezione ambientale, negli articoli 6, 10 e 11, una serie di funzioni di indirizzo e coordinamento dell'intero Sistema nazionale, lasciando all'ISPRA il compito di individuare le linee di intervento per assicurare il raggiungimento dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) su tutto il territorio nazionale. L'Istituto assume poi la responsabilità di provvedere alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale, cosa ancora più importante, se si considera che il disegno di legge prevede, per tutti gli enti locali e per tutte le associazioni ambientaliste legalmente riconosciute, la fruizione libera dei dati e addirittura la possibilità di avanzare richieste su specifici valori ambientali. Ora, tutto l'impianto del disegno di legge è evidentemente improntato a un disegno armonico di coordinamento e di maggiore efficacia della rete del Sistema nazionale di protezione ambientale. Il problema però è capire se questo nuovo Sistema possa funzionare. E il primo grande dubbio sorge leggendo il nuovo articolo 17, inserito dalla Commissione alla Camera, che prevede l'obbligo di invarianza finanziaria per tutto il disegno di legge. Ci si chiede se, sempre rispettosi comunque delle finanze pubbliche, una riorganizzazione così complessa e radicale di un settore nevralgico per il nostro Paese possa essere fatta a costo zero, senza prevedere neanche uno sforzo economico iniziale. Temiamo, quindi, di trovarci di fronte al solito gioco di prestigio del primo ministro Renzi: una bella narrazione, efficace e convincente, a cui seguono inevitabilmente provvedimenti legislativi deboli, inutili, sbagliati o totalmente inefficaci; una manipolazione continua della realtà, per cui il Paese riparte, ma non si muove; gli occupati aumentano e poi si scopre che non è vero; il PIL si impenna, ma poi effettivamente

Da quello che so, il concetto stesso di rete implica l'orizzontalità, la sostanziale equivalenza di tutte le componenti. Qui invece viene costruita, più che una rete, una piramide, al cui vertice c'è l'ISPRA, che, seppure posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, risulterà essere il vero *dominus* della questione ambientale; insomma, una sorta di mano armata di qualunque Governo, che sarà in grado di dettare la politica ambientale del nostro Paese, con scarsissimi controlli terzi e *super partes*. Infine, vorrei sottolineare come con questa riforma di impronta fortemente centralista si rischia di appiattire in un unico standard minimo le eccellenze che, in questi anni, si sono formate a livello di ricerca, di strumenti contro gli abusi ambientali, di prevenzione dei danni alla salute pubblica e in molti altri campi ancora. C'è insomma il rischio che il sistema dei LEPTA, coordinato e controllato dall'ISPRA, riduca le varie Agenzie regionali a occuparsi solo ed esclusivamente dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di ambiente. E questo sarebbe un danno per tutte quelle realtà che, in varie parti d'Italia, in questi anni hanno sviluppato professionalità e modalità di intervento di altissima qualità. Non posso che concludere quindi, con mio sommo rammarico, che anche in questo caso si tratta di un'occasione persa. persa. È vero che le Agenzie regionali avevano bisogno di una nuova sistemazione organica e che l'ISPRA da tempo aspettava una nuova personalità giuridica, con nuove funzioni e responsabilità. Ma il nostro ambiente avrebbe meritato uno sforzo maggiore e risultati migliori di quelli che porterà questo inutile, se non dannoso, disegno legge. *(Applausi del

il disegno di legge in esame ha per oggetto un tema di particolare rilevanza per un Paese che vuole perseguire un livello sempre più alto di tutela dell'ambiente, ovvero l'istituzione di un Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è stato istituito

e comprende norme che istituiscono e disciplinano il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Le funzioni dell'ISPRA ricomprendono, tra l'altro, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali. Queste ultime costituiscono standard qualitativi equantitativi di attività che devono essere garantite in modo omogeneo a livello nazionale e rappresentano il parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie, al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale. A quest'ultimo viene affidata, tra le altre cose, un'articolata serie di funzioni di indirizzo, coordinamento tecnico, controllo, monitoraggio, ricerca, consulenza tecnica e formazione.

Il relativo provvedimento, tra l'altro, risale al 1994. Come Gruppo della Lega Nord, oltre a mettere in condizione la maggioranza di poter esaminare degli emendamenti certamente

per garantire un'articolata, ma omogenea disciplina per le attività dell'ARPA, ponendo fine alla situazione attualmente esistente nelle diverse aree del Paese, le quali, seppur con con idee e leggi abbastanza simili, chiaramente non avevano la possibilità, se non in alcuni punti, di interagire tra di loro.

quella che veniva considerata alcuni anni fa a scuola l'educazione civica, che potrebbe mettere in condizione il nostro Paese di essere veramente "il bel Paese". Siamo dunque d'accordo che esistono aspetti del Sistema delle Agenzie che occorre riorganizzare e razionalizzare, anche se temiamo che la revisione della normativa vigente debba avvenire in rapporto alle normative regionali regionali di riferimento per le singole Agenzie regionali, lasciando sempre la Regione come organo di vigilanza sulla singola Agenzia. Qui mi verrebbe da fare una chiosa: se non dovesse passare il*referendum*,

pertanto il provvedimento utile per restituire credibilità tra i cittadini sul sistema dei controlli ambientali e riaccendere la fiducia della popolazione verso le istituzioni, attraverso attraverso l'applicazione di norme certe e limiti ambientali omogenei su tutto il territorio. E, quando parlo di tutto il territorio, chiaramente faccio riferimento a quanto dicevo prima: rivolgere un'attenzione alle problematiche ambientali che abbia la stessa omogeneità

il provvedimento in Commissione e di valutarlo sotto tutti gli aspetti, chiaramente ha messo in luce alcune

Uno dei punti principali sarebbe stato il finanziamento del Sistema. Si dice sempre che senza soldi non si cantano messe, e questo vale anche per l'ISPRA. Il testo attuale ha congelato il problema del finanziamento delle ARPA, mentre questo, in analogia al finanziamento del Sistema sanitario nazionale, come già apparso apparso nelle prime bozze del progetto di legge alla Camera, rappresenta un punto fondamentale per una vera riforma dell'intero Sistema. è la convivenza tra la natura di istituto di ricerca dell'ISPRA e i nuovi compiti di coordinamento delle Agenzie regionali di attività di monitoraggio. La nuova legge interviene sui compiti di ricerca dell'ISPRA, lasciando invariata la normativa vigente, ma senz'altro, l'accavallamento delle competenze potrebbe creare problemi

assicura il passaggio delle informazioni e la collaborazione tra le Agenzie, l'ISPRA e gli altri enti di ricerca, determina economie di gestione, soddisfa una sempre più cogente le necessità dei cittadini di riconoscere questi istituti questi istituti a tutela dell'ambiente in cui viviamo e le potenzialità di sviluppo. Pensiamo che sicuramente si sarebbe potuto fare meglio in questo provvedimento. La questione legata all'ambiente è parte

per dotarsi di un Sistema nazionale di protezione dell'ambiente, che veramente risponda alle esigenze dei nostri tempi e alla domanda di salute e di sicurezza ambientale rivoltaci dai cittadini. Alla luce delle numerose problematiche che affliggono l'Italia su questo controverso fronte, è emerso più volte come in passato la separazione delle competenze sanitarie e ambientali, da un lato, abbia focalizzato l'attenzione sulla tutela dell'ecosistema e sui suoi fragili equilibri, ma dall'altro, abbia probabilmente lasciato la salute dei cittadini relativamente scoperta rispetto all'impatto delle attività, siano esse lecite o illecite. Così, il bilancio delle politiche ambientali italiane per la tutela della salute si è rivelato spesso largamente insufficiente, come provato da alcuni casi eclatanti come la diossina in Campania, il caso ILVA, l'arsenico nelle acque e le crescenti paure della popolazione, che sfociano in quella che è stata battezzata la sindrome NIMBY. Le imprese si lamentano dell'eccessiva burocrazia richiesta dalle pratiche ambientali; ASL e Agenzie ambientali regionali spesso non lavorano in sinergia e sono ancora troppi i pregiudizi e le ideologie, con la conseguenza che spesso i cittadini lamentano di non sentirsi sufficientemente tutelati dai fattori ambientali lesivi della salute umana. Non sono rari, infatti, i casi in cui, pur in assenza di specifiche violazioni delle leggi ambientali, si determina comunque un danno alla salute dei cittadini. Ben venga quindi, in questo quadro, un provvedimento che valorizzi e metta a sistema quelle competenze specialistiche dedicate ai controlli ambientali che, dal 1993 in poi, sono state costruite e dia stessi controlli ambientali una forza maggiore. Infatti, in questi anni, si è proceduto a macchia di leopardo: in alcune Regioni Agenzie regionali costituiscono delle strutture di eccellenza, mentre in altre Regioni il funzionamento è nettamente peggiore; inoltre non tutte le Agenzie regionali godono di certezza di finanziamenti, e questo costituisce un serio problema. Oggi, poiché ambiente e salute stanno razionalmente insieme e oramai è pacifico che si debbano superare tutte le difficoltà interpretative che possono aver portato la Sanità quasi a disinteressarsi delle questioni ambientali, non possiamo che guardare con fiducia a questa riforma, che conferma lo sforzo di omogeneizzare le attività delle Agenzie di protezione dell'ambiente sparse nel territorio nazionale e di configurare con chiarezza i ruoli e le funzioni di ISPRA. Riteniamo, infatti, che l'aspetto più qualificante del provvedimento sia quello di aver avvistato nei LEPTA, cioè i livelli essenziali di tutela ambientale, il minimo comune denominatore per tutte le Agenzie regionali. Si tratta di un Sistema che interagisce con la Sanità e con i LEA (livelli essenziali di assistenza sanitaria), per garantire il perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva; un sistema che costituirà un livello uniforme in tutto il territorio nazionale per le attività di monitoraggio, controllo, ricerca finalizzata, sviluppo delle conoscenze e diffusione dei dati tecnico-scientifici, supporto tecnico-scientifico. Veramente questo nuovo Sistema nazionale può rappresentare una svolta e un salto di qualità, non dimenticando però mai il contenimento della spesa e un'applicazione più pregnante del principio del «chi inquina paga». Pertanto, dal nostro punto di vista, l'approvazione di questo provvedimento è non solo importante, ma anche necessaria, per permetterci di lavorare con una migliore qualità; per consentirci di raccogliere una sfida importante di protezione dell'ambiente, ma soprattutto per cementare una relazione tra ambiente e salute, che deve essere oltremodo rinsaldata non solo nella politica e nell'amministrazione, ma anche nel tessuto produttivo del nostro Paese. Le problematiche ambientali , infatti sono trasversali e rilevanti in ogni settore della vita. Di questo i cittadini si sono accorti già da tempo e ci chiedono di prestare sempre più attenzione alla salute dell'ambiente, che inevitabilmente diventa salute per l'essere umano e che sempre più diventerà domanda di sicurezza alimentare e di protezione dell'ambiente agricolo. Ben venga quindi questo provvedimento. Ben vengano tutte le misure di modernizzazione di un Sistema di protezione ambientale che, troppo spesso e troppo a lungo, ha scontato uno stato di inadeguatezza e di arretratezza legislativa, a cui oggi abbiamo l'occasione di porre fine. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame ha a oggetto un tema di particolare rilevanza in un Paese che sta lavorando per un livello sempre più alto di tutela dell'ambiente. L'istituzione di un Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente non solo è finalizzato ad armonizzare, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, le attività delle Agenzie sul territorio, le ARPA, ma soprattutto realizza un sistema integrato di controlli coordinati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Storicamente, prima con la legge n. 61 del 21 gennaio 1994 (istituzione Agenzia nazionale protezione ambientale) e successivamente col decreto-legge n. 112 del 2008 2008 (istituzione dell'ISPRA), le Agenzie per la protezione ambientale hanno sempre rappresentato il soggetto istituzionale competente e di riferimento a livello locale per tutte le questioni in materia ambientale. Inoltre, le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale, di prevenzione, controllo e vigilanza finalizzate alla protezione dell'ambiente sono state integrate con funzioni di consulenza e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni nonché agli enti pubblici. Vale la pena ricordare, per l'appunto, che le Agenzie sono state istituite al fine di rispondere in modo adeguato e tempestivo alle istanze esterne, sia per quanto riguarda gli eventi a impatto ambientale sia con riferimento alla ricca normativa di riferimento Quindi, le funzioni svolte - indubbiamente di natura pubblica - riconducono l'applicazione sistematica di conoscenze tecniche e scientifiche organizzate al fine di supportare e implementare le politiche regionali in materia di ambiente. Nondimeno, il quadro istituzionale di riferimento individua, quali principali interlocutori di riferimento, i soggetti pubblici e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali. Entrando nel merito delle disposizioni contenute nel disegno di legge che andiamo ad approvare, mi trovo particolarmente concorde con la riorganizzazione della struttura, coordinata a livello centrale e armonizzata a livello regionale. Certo, la clausola di invarianza finanziaria, inserita ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ci ricorda che il momento attuale impone alle pubbliche amministrazioni di essere improntate all'efficienza, all'efficacia, ma soprattutto al contenimento dei costi. Sicuramente, il nuovo metodo che si verrà a creare per gestire e pianificare l'azione pubblica in materia ambientale - che, ricordo a tutti, andrebbe inteso sempre più come prevenzione e sempre meno come risposta alla emergenza - dovrà essere un concreto supporto tecnico-scientifico, assicurato dalla rete delle Agenzie e dall'ISPRA, che svolgerà ricerche, monitoraggi, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente e del territorio. In questa direzione si colloca la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal sistema nazionale al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali. Un altro punto di seria riflessione è, poi, quello di una gestione sempre più sostenibile del territorio e delle sue risorse. e di gestione eco-compatibile del territorio, non basta solo un'integrazione della normativa nazionale con quella comunitaria, ma occorre anche una diffusa presa di coscienza del rispetto del territorio, delle sue caratteristiche e della prevenzione dei rischi in cui può incorrere. incorrere. La spinta propulsiva, infatti, che hanno dato soprattutto le normative comunitarie ha profondamente modificato il diritto ambientale e riformato l'amministrazione pubblica, riconoscendo, al contempo, il ruolo fondamentale delle politiche ambientali nello sviluppo economico del Paese. Paese. Approvo con molta soddisfazione anche l'impostazione data al nuovo Sistema nazionale di protezione ambientale introdotto da questo provvedimento: esso svolgerà un autonomo ruolo, un ruolo tecnico-scientifico e non più solamente operativo delle amministrazioni pubbliche, alle quali era ricondotta la vigilanza. A dire il vero, anche il ruolo operativo di vigilanza è stato potenziato con l'acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria da parte del personale, prevedendo che a tale personale siano garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. Questo comporterà maggiori responsabilità nella gestione, pur restando comunque sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto riguarda l'ISPRA, e delle Regioni, per quanto riguarda invece le ARPA. Concludendo, il mio personale giudizio è certamente positivo, confermando un ulteriore passo avanti, con questo disegno di legge, dopo l'introduzione, lo scorso anno, della legge n. 68 sui reati ambientali, verso la comprensione e la risoluzione dei complessi problemi legati all'ambiente. Tutto questo non basta probabilmente, aspettiamo di compiere altri passi come, ad esempio, il disegno di legge sul consumo di suolo o una nuova normativa sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. La ottimale gestione del territorio rappresenta la sfida per l'eccellenza futura: procediamo su questa strada.

È proprio per questo motivo che la Commissione 13a al Senato non ha voluto apportare alcuna modifica al testo licenziato dalla Camera, tranne l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria della quale sinceramente, a nostro parere, non c'era esplicitamente bisogno, ma che, in ottemperanza ai Regolamenti e anche alla legge, siamo stati costretti ad inserire.

che vide l'83 per cento degli italiani votare «sì» riguardo all'ipotesi di enucleare le mansioni di controllo sull'ambiente dalle strutture delle organizzazioni sanitarie al fine di esaltarne la specificità e, quindi, con la consapevolezza di quanto fosse importante, già a quel tempo, un controllo reale sull'ambiente, con tutte le implicazioni che derivano e derivarono da quella intuizione. è precisamente da quel momento che ha avuto inizio un percorso di natura normativa, organizzativa ed operativa a conclusione del quale si è costituito un sistema di Agenzie,

A seguito degli esiti del *referendum*, fu promulgata la legge n. 61 del 1994, che conteneva disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli ambientali, sull'istituzione dell'Agenzia nazionale e indicava anche che Regioni e Province autonome si dotassero, attraverso proprie leggi, di Agenzie regionali. Le leggi regionali sono state promulgate in un arco temporale piuttosto lungo, durato circa dieci anni, fino al 2006 e per molte Agenzie e Regioni, dopo la prima legge istitutiva, vi sono già stati significativi aggiornamenti normativi. Ma bisogna riconoscere come ciascuna Regione, nella propria autonomia, ha lavorato e legiferato in maniera diversa, istituendola propria Agenzia ambientale,

non solo una disomogeneità teorica sul territorio nazionale, ma anche una certa distonia che, in un certo qual modo, crea difficoltà a cittadini e imprese. Basti pensare a grandi imprese, che lavorano su tutto il territorio nazionale che si trovano a impattare, Regione per Regione, con regolamenti, procedure e *iter* procedimentali completamente diversi l'uno dall'altro. È altrettanto vero, però, che le problematiche operative, che costituiscono il fulcro di quasi tutte le Agenzie, e i controlli sulle fonti di emissione e i monitoraggi sullo stato dell'ambiente presentano, viceversa, problematicità omogenee a cui bisogna dare risposte univoche, qualsiasi sia il territorio dove vivono i cittadini. Vi sono, dunque, alcuni aspetti del complesso lavoro di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema che dovranno essere chiariti, a partire dalla necessità di garantire una definizione di sistema agenziale che oggi non può che essere un sistema organizzativo in grado di dare risposte tecniche efficaci a costi minimizzati. Le attese più forti sono sul cambiamento e sulla stabilizzazione del ruolo e delle funzioni delle Agenzie ambientali, ruolo ruolo che deve cambiare perché oggi sta cambiando il modo di essere della pubblica amministrazione. Deve cambiare poiché deve consolidare l'importante aspetto tecnico di ciascuna Agenzia a supporto della prevenzione sanitaria e ambientale; deve cambiare poiché la sensibilità dei cittadini, nelle materie ambientali e di prevenzione ambientali e di prevenzione della salute collettiva, intesa come bene primario da tutelare, è sempre crescente e ha bisogno di risposte chiare e trasparenti, oltre che tecnicamente ineccepibili. Pertanto, l'articolato del disegno di legge provvede all'istituzione di un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (il cosiddetto Sistema nazionale), di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente,

della riforma costituzionale, che ha voluto inserire proprio l'ambiente tra i beni sottoposti a tutela costituzionale come interesse primario per il Paese. Il Sistema nazionale ha una pluralità di compiti ben definiti, tra cui il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione, il controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle "pressioni sull'ambiente", l'attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale, il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, la partecipazione ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché la collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione, l'attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali, le funzioni

di trasferire all'ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino. Si attribuisce inoltre alle Agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le Agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali nei rispettivi territori di competenza. Credo che questo sia un concetto fondamentale, perché proprio questi livelli essenziali costituiscono quel livello minimo omogeneo che deve valere su tutto il territorio nazionale che il Sistema nazionale è pertanto tenuto a garantire, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. L'ISPRA dovrà infatti programmare le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento di questi livelli essenziali sull'intero territorio nazionale e garantire l'approvazione del programma che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani e delle attività delle singole Agenzie. Al fine di uniformare a livello nazionale le modalità di analisi dei dati, si è ritenuta opportuna la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale, al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali. Il Sistema nazionale è - sì - tenuto a ricorrere in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni, ma, sapendo quanto sia notevole la mole di lavoro, ha anche la possibilità possibilità di rivolgersi, alla bisogna, ai laboratori esterni, che devono però rispondere a quei criteri di omogeneità che, come ho detto, valgono su tutto il territorio nazionale Per finanziare l'attività dell'ISPRA si prevede la concessione di un contributo statale che si configura come integrativo rispetto alla dotazione ordinaria, quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività. Tutto questo consente all'ISPRA e alle Agenzie l'assunzione di personale e l'acquisizione di beni strumentali per le finalità della legge e nei limiti delle risorse finanziarie indicate. Appare evidente, quindi, che la strada che il disegno di legge in esame intende percorrere è quella di un'uniformità di mansioni da compiere in trasparenza e nel raggiungimento di un

cercando di capire e intuire quali siano i settori della ricerca che non ha più senso che stiano dentro l'ISPRA o il Sistema nazionale delle Agenzie e debbano confluire in un grande sistema della ricerca pubblica, che può essere garantito dalle università

sia conoscitiva, che di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche indispensabili di sostenibilità. È un dato di fatto come 21 Agenzie abbiano portato in evidenza in questi anni che ruoli e risorse differenziate e assolutamente non omogenee hanno di fatto impedito che la qualità ambientale potesse essere istituita a sistema Paese, con una convergenza di strategie operative e di modalità di esercizio nei compiti istituzionali. Si è quindi generata incertezza per le aziende e per i cittadini, ma anche perplessità, incertezza e incoerenza per le stesse realtà istituzionali comunali e per gli operatori economici.

nonché degli stessi costi *standard*, ma direi che è un passo avanti di straordinaria chiarezza e trasparenza; insomma, viene messo nero su bianco il livello della qualità di aria, suolo e acqua cui hanno diritto i cittadini italiani. quindi che questo proceda nella salvaguardia della biodiversità, nei monitoraggi corretti per i cambiamenti climatici, nella verifica del dissesto idrogeologico.

ci sia una rete omogenea, che si muove in maniera pressoché omogenea in tutto il territorio nazionale, rende davvero possibile pensare a un futuro molto diverso rispetto al passato.

del territorio e del mare, l'ISPRA e il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, oltre che per le stesse ARPA. Abbiamo da sempre sostenuto che per portare avanti con successo il tema del rispetto ambientale per uno sviluppo sostenibile è necessario un gioco di squadra, che metta in sinergia e a frutto tutte le capacità che abbiamo.

di opacità di questo disegno di legge e che speriamo di sanare in tempi rapidi: non si può immaginare di fotografare una realtà disomogenea trasformandola in omogenea senza prevedere, inevitabilmente, un un livello legislativo che produca un'azione di livellamento e quindi di qualità tale per cui tutte le Agenzie locali siano messe sullo stesso piano, o un intervento economico da parte dello Stato,

Signora Presidente, prima di entrare nel merito del provvedimento di cui discutiamo, vorrei soffermarmi su di un fatto che è stato fondamentale per il sistema agenziale: mi riferisco al *referendum* abrogativo del 1993, con il quale i cittadini hanno chiaramente manifestato la volontà di sottrarre al Servizio sanitario le competenze in materia di protezione ambientale al fine di garantire una maggiore autonomia alle Agenzie. Questo è un dato particolarmente rilevante non solo perché da quel momento in poi si è costituito effettivamente il sistema delle Agenzie ambientali, ma soprattutto perché rappresenta uno dei pochissimi casi in cui si è dato seguito alla volontà popolare, evento anomalo per i Governi che si sono susseguiti negli ultimi anni. Lo sa bene il Governo Renzi, che non solo non tiene in considerazione la volontà referendaria espressa nel 2011 da 26 milioni di italiani relativamente alla gestione dell'acqua pubblica, ma anzi si spinge oltre. Come sapete tutti bene, in modo palese questo Governo sta calpestando il diritto e dovere di voto dei cittadini: in occasione dell'ultimo *referendum* sulle trivelle Renzi ha invitato i cittadini a non andare a votare, solo per favorire le *lobby* dei petrolieri. Secondo il nostro punto di vista questo è inaccettabile. Ma torniamo alle Agenzie. Il disegno di legge di cui discutiamo oggi è il frutto di un lavoro di coordinamento che è stato svolto anche grazie al Movimento 5 Stelle, considerato che uno dei disegni di legge è a prima firma del collega Massimo De Rosa, così come già successo per il disegno di legge sui reati ambientali. Tale lavoro congiunto è stato possibile però solo alla Camera, considerato che qui in Senato non ci è stata data l'opportunità di intervenire con puntuali proposte (tutti gli emendamenti, in Commissione, hanno ricevuto parere contrario) ed è da rilevare che il provvedimento è stato parcheggiato in Commissione ambiente da aprile 2014. C'è stato un vero e proprio ostruzionismo da parte del Governo, che evidentemente non digerisce questo testo e ha cercato di bloccarlo in tutti i modi. Eppure, in Commissione non vi è stata una contrapposizione fra i vari Gruppi politici, ma solo da parte del Governo che, come fa ormai spesso, si è intromesso con forza nell'ordinaria attività parlamentare. Avevamo deciso, infatti, con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, al solo scopo di agevolare la conclusione dei lavori, di non apportare alcun ulteriore cambiamento al testo, ma di limitarci alla presentazione di ordini del giorno. Ma fino alla fine abbiamo dovuto subire l'ennesimo atto di prepotenza, con l'emendamento del relatore dell'ultimo minuto, non emendabile, scritto su richiesta della Ragioneria di Stato che, guarda caso, dopo un anno ha cambiato idea, inserendo una clausola di invarianza economica su tutto il provvedimento. legge sulle Agenzie dovrebbe essere considerato come il giusto completamento del disegno di legge sugli ecoreati. In effetti, che senso ha prevedere sanzioni per i reati ambientali se poi non si può contare su un'attività di controllo coordinato sul territorio necessaria per la tutela ambientale? Non posso in tale contesto non denunciare che il sistema di protezione dell'ambiente progettato, non potrà contare sul valido supporto tecnico del Corpo forestale. Il sistema di coordinamento ambientale, infatti, non si concilia con l'assurda decisione del Governo di sopprimere il Corpo forestale dello Stato, l'unico corpo di polizia da sempre impegnato in materia ambientale, il cui ruolo speciale e specialistico è ormai in modo definitivo compromesso con l'accorpamento nell'Arma dei carabinieri. Nelle nostre intenzioni ARPA e ISPRA devono diventare enti che stanno dalla parte del cittadino, che agiscono per tutelare la salute, l'ambiente e il territorio, il vero patrimonio dello Stato. Anche per questo abbiamo proposto, con un ordine del giorno, che a coloro che esercitano funzioni ispettive venga riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, andando tra l'altro a porre fine ad una discriminazione che si verifica tra le varie Agenzie regionali. Oggi, infatti, a macchia di leopardo alcune ARPA riconoscono tale qualifica a tutti coloro che svolgono funzioni ispettive. È necessario, quindi, un intervento specifico onde evitare diseguaglianze. Devo segnalare che alcuni punti, che riteniamo particolarmente rilevanti, non sono stati accolti: avremmo voluto Agenzie più indipendenti e autonome, che svolgessero controlli anche sulle scelte politiche in materia di ambiente, analizzando dal punto di vista tecnico le conseguenze sul territorio delle scelte fatte in questi Palazzi. Purtroppo, non siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi perché è mancato l'appoggio della maggioranza, ma abbiamo migliorato di molto il testo. Ad esempio, abbiamo introdotto dei vincoli per cui le figure, come i direttori generali e i presidenti, debbano essere necessariamente figure di rilievo per competenza tecnico-scientifica e prive di conflitti con altre cariche. Abbiamo, anche in tale contesto, detto no alla casta e alle scelte imposte dall'alto, puntando sul merito e sulle competenze. Inoltre, abbiamo inserito degli indirizzi per far tendere il sistema delle Agenzie ai massimi *standard* tecnico-scientifici internazionali. In questo modo, i tecnici tenuti al monitoraggio lo faranno con i sistemi più all'avanguardia e più efficaci che ci siano, con *standard* che, tra l'altro, saranno soggetti ad un adeguamento costante in base alle eventuali criticità ambientali emerse. Altra caratteristica a «5 Stelle» che si rintraccia nel disegno di legge è la creazione di un *database* di dati ambientali accessibile, in modo che i dati ambientali siano trasparenti e fruibili a chiunque, soprattutto ai semplici cittadini, che riscontrano molte difficoltà burocratiche. Al di là del contenuto, permettetemi, infine, di fare una riflessione sulle modalità di attuazione della disciplina. La maggior parte degli articoli rinvia infatti a successivi decreti attuativi, problema evidenziato non solo da noi ma anche da vari soggetti auditi in Commissione, come ad esempio la AssoArpa, che ha rilevato il fatto che il provvedimento, non essendo *self-executing*, può generare non poche incertezze e ritardi applicativi. Considerato che siamo abituati non solo ai ritardi ma molto spesso alle inadempienze amministrative, abbiamo presentato al proposito un emendamento ed anche un ordine del giorno, con i quali proponiamo di inserire un apposito sistema sanzionatorio collegato al ciclo delle *performance*, in modo che il soggetto responsabile dell'adozione dell'atto amministrativo possa essere maggiormente responsabilizzato, anche con eventuali sanzioni disciplinari. Altra questione particolarmente delicata è il finanziamento delle Agenzie. È chiaro che se non si prevedono risorse adeguate, ogni fonte di entrata può andare a compromettere l'indipendenza del sistema delle Agenzie. Per questo motivo, avevamo proposto che venisse disposta la garanzia di un finanziamento imparziale, destinando, quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente. Inutile dirvi che non ci avete ascoltato. Il Movimento 5 Stelle ha proposto altresì la creazione di un apposito fondo ambientale, nell'ambito del Fondo unico giustizia, finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, destinato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati. Come ho già anticipato, nell'ultimo giorno di esame del provvedimento in Commissione ambiente è arrivato l'emendamento suggerito dalla Ragioneria sull'invarianza economica. Le risorse previste erano già risicate, se non vi devono essere ulteriori oneri, come faranno ad esercitare le loro funzioni queste Agenzie? Significa che diventa un provvedimento di facciata e che, all'atto pratico, non vi è la possibilità di lavorare concretamente. Non si comprende, inoltre, come mai la Ragioneria faccia una valutazione diversa da quella fatta alla Camera e perché abbia impiegato un anno per farla. La verità è che si tratta solo di un altro tentativo di impantanare il provvedimento. Infatti ora, con questo nuovo intervento modificativo, il testo dovrà tornare nuovamente all'esame della Camera, spero per non essere nuovamente insabbiato. Concludendo, sono trascorsi ormai due anni da quando questo provvedimento è stato incardinato in Commissione ambiente in Senato, ed è stato tenuto fermo in attesa che il Governo decidesse quando e come portarlo in Aula. Eppure, questo disegno di legge aveva incontrato il favore della maggioranza dei Gruppi politici. Certo, si poteva ulteriormente migliorare, ma quantomeno poteva essere votato già da tempo, se non fossimo stati costretti a sottostare ai capricci di un Governo che si mette sempre di traverso, dimenticandosi che il potere legislativo è ancora nelle mani delle Camere e che il Governo dovrebbe semplicemente essere un organo "esecutivo". Ma ormai siamo ben consci dello stato dittatoriale nel quale siamo caduti e di cui sicuramente ci libereremo presto. Nel frattempo, ci auguriamo che questo provvedimento riesca a passare, almeno così com'è.

Purtuttavia, non posso non esprimere alcune preoccupazioni. Partendo dalla coda, la prima preoccupazione è

finanziaria, perché, da che mondo è mondo, non si ristrutturano i Ministeri e non si introducono nuove Agenzie e nuovi organi collegiali senza provvedere minimamente a spendere un po' di denari. Quindi, ancora una volta, ci si trincera dietro una clausola di invarianza finanziaria che è solamente un'indicazione formale. Da questo punto di vista, d'accordo con il Presidente della Commissione bilancio e con gli altri Gruppi, presto avvieremo un un affare assegnato, come si dice in gergo parlamentare, per controllare se tutte queste clausole grazie alle quali passano le leggi, perché vengono esentate dalla censura dell'articolo 81,

perché, se è vero che cose nuove si possono fare con gli stessi stanziamenti, questo allora significa che nei Ministeri ci sono degli sprechi. Il presupposto che questo non comporti un aggravio di spesa significa che le cose che si facevano prima venivano fatte con somme esorbitanti rispetto alle necessità, dato che ci sono, nei capitoli di bilancio, spazi per poter assolvere

purtroppo, molto spesso i rendiconti sono la cosa che in questo Parlamento passano nella maniera più veloce e più acritica, rispetto a tanti altri provvedimenti, mentre dovrebbero essere veramente analizzati dal Parlamento. Detto

a dire la verità; essi cercano invece di arrampicarsi sugli specchi, per avallare alcune scelte governative. L'ultimo caso emblematico, che è stato già ricordato, è stato quello di alcune valutazioni

stati resi in maniera molto più politica che non tecnica (mi limito a questa piccola osservazione). Quindi questo provvedimento, che vuole mettere ordine e che reintroduce una sorta di regia centrale su quella che veniva ritenuta un'eccessiva frammentazione, alle volte anche contraddittoria, tra un ente regionale e l'altro, spero e vorrei che non sia un tentativo di normalizzazione, anche dal punto di vista di un'attività di controllo e di un'attività di intervento che deve essere assolutamente e ferreamente efficiente e soprattutto organizzata su criteri di verità scientifica e non su criteri di esigenza politica. Questo è quello che noi temiamo dal punto di vista del rapporto, che diventa sempre più di dipendenza, tra autorità politica e organismo tecnico. Questo ci preoccupa, perché nel nostro Paese esistono enormi varietà di situazioni dal punto vista ambientale. Qui si tende non tanto e non solo a razionalizzare, che potrebbe anche essere giustificabile, ma si tende anche ad omogeneizzare, su scala nazionale, alcune valutazioni che invece dovrebbero trovare non tanto nella dimensione regionale, dal punto di vista amministrativo dal punto di vista amministrativo o geografico, ma nella dimensione locale la valutazione di alcune caratteristiche che sono assolutamente differenti tra un punto e l'altro del nostro Paese. Noi abbiamo chiesto che l'attività dell'ISPRA e dell'Agenzia diventi supporto non solamente dei livelli nazionali e regionali, ma anche dei livelli comunali. Credo che l'emendamento non sarà approvato, perché l'indirizzo è quello di varare il testo nella formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati e quindi di renderne definitiva la lettura, tranne che per l'articolo 17, che poi andrà alla Camera ‑ immagino ‑ per una rapida ratifica. Abbiamo chiesto questo perché riteniamo che, con i tempi che corrono, soprattutto di esigenze della finanza locale, un'Agenzia nazionale possa essere effettivamente di supporto ai Comuni nelle loro esigenze. Recentemente abbiamo assistito a una vicenda incredibile:

È assolutamente indescrivibile quello che sta accadendo nei rapporti tra gli enti locali il Governo: un Comune, che già dovrebbe chiedere miliardi di danni dal punto di vista ambientale per il ripristino di zone straordinariamente belle e dalle straordinarie potenzialità

l'infrazione comunitaria dovuta all'inquinamento, per scelte assolutamente disastrose dal punto di vista ambientale - ma io dico, anche dal punto di vista sociale, industriale ed economico - fatte non certo da quel Comune. Comune. Non sono stati certamente i Comuni di Augusta e Priolo, infatti, a chiedere l'insediamento delle raffinerie e delle strutture industriali inquinanti sul proprio territorio.

tace, quando deve imporre a determinati soggetti di ripristinare l'ambiente spendendo le somme che è giusto spendere perché questo ambiente venga ripristinato.

essa non segni un passaggio alla normalizzazione degli indirizzi governativi di organismi tecnici, che non dovrebbero essere assolutamente non influenzati dagli indirizzi governativi e soprattutto dovrebbero difendere lo straordinario patrimonio di paesaggio e di ambiente del nostro Paese. PRESIDENTE. Signora Presidente, onorevoli colleghi, cara Sottosegretaria, il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi nasce da molto lontano. È una riforma su cui si discute da almeno otto anni e che, a due anni dalla sua approvazione alla Camera, per una modifica tecnica che non siamo riusciti ad evitare di inserire, stiamo rimandando alla Camera per la sua terza e, mi auguro, Come Partito Democratico e come Governo abbiamo messo in campo, durante questa legislatura, un pacchetto di norme per una vera e propria riforma ambientale che nel garantire maggiori tutele per l'ambiente favorisca il reale sviluppo della *green economy* nel nostro Paese. Perché la tutela dell'ambiente non è solo un imperativo morale, ma è soprattutto l'occasione per promuovere finalmente l'imprenditoria sana, quella che soffre la concorrenza di quanti operano nella zona grigia, ricorrendo all'illecito ambientale per risparmiare. L'approvazione di questo disegno di legge, che riordina il sistema delle Agenzie ambientali, si rende quindi fondamentale per dare piena attuazione alle misure contenute nella legge sugli ecoreati e nel collegato ambiente, restituendo indipendenza e professionalità ai tecnici specializzati nella tutela ambientale, nonché contribuendo a riequilibrare le differenze tra le varie Regioni e a recuperare le situazioni di maggiore ritardo. Non dobbiamo dimenticare, colleghi, che le domande e le preoccupazioni dei cittadini riguardo al tema della tutela ambientale e dei rischi per la salute richiedono da tempo una risposta da parte delle istituzioni, che sia credibile credibile e al passo con i tempi. Da quando è iniziata questa legislatura numerosi sono stati i provvedimenti varati d'urgenza per limitare i danni ambientali e alla salute: ora è necessario cambiare paradigma, fornire nuove risposte, restituendo ad esempio agli organi tecnici preposti ai controlli quell'autorevolezza indispensabile per far sentire i cittadini tutelati nel bene supremo che è la propria salute. La costruzione di un sistema di Agenzie di protezione ambientale, che garantisca conoscenza, trasparenza e professionalità diventa, quindi, una priorità assoluta. La loro costituzione, con la legge n. n. 61 del 1994, ha segnato un traguardo importante, ma ora è necessario andare oltre. Sicuramente non partiamo da zero. Già oggi le Agenzie e contano oltre duecento sedi al servizio del Paese, 600.000 campioni analizzati ogni anno, quasi 100.000 operazioni tra ispezioni e sopralluoghi, oltre 73.000 istruttorie e pareri, più di 11.000 operatori coinvolti. Si tratta di numeri importanti, numeri importanti, ma che non garantiscono un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei controlli necessari. Le Agenzie del Sud sono sicuramente le più in difficoltà,

Con questo provvedimento si dà finalmente al Paese un'organizzazione efficace ed efficiente del sistema dei controlli. Non si tratta solo di verificare il rispetto delle norme, di assoluta importanza, ma di articolare e regolamentare anche quella complessa attività di monitoraggio e raccolta dati, che serve per migliorare il grado di conoscenza dei numerosi fattori ambientali. In questo modo il decisore politico - cioè noi - potrà avere a disposizione dati certi, scientificamente validati, prodotti da organismi tecnici autonomi, che gli consentiranno di decidere in modo consapevole per il bene delle nostre comunità. Vedete colleghi, ogni qual volta nel nostro Paese si prova a parlare della necessità di costruire un qualsiasi tipo di impianto o infrastruttura, si manifestano pesanti fenomeni di conflittualità sociale, di conflittualità sociale, spesso dovuta alla scarsa fiducia dei cittadini verso le istituzioni politiche e amministrative, ma anche verso quelle tecniche, sempre più accusate di essere asservite alle decisioni della politica, se non - peggio - a quelle del malaffare. Il provvedimento che andiamo a votare, quindi, contiene misure che, nel fornire più più autonomia alle Agenzie e all'ISPRA, definiscono in maniera chiara il rapporto fra controllore e controllato, chiedono più professionalità a chi dovrà dirigere queste organizzazioni che, pur rimanendo strutture tecniche strumentali, formuleranno pareri, che saranno vincolanti per le autorità competenti. Si costruisce un vero e proprio sistema a rete, coordinato dall'ISPRA. Rimane però la completa autonomia dei livelli regionali e si realizzano sinergie fra gli enti, mettendo in rete numerosi laboratori provinciali. In questo modo si determinano dei livelli di prestazione tecnica ambientale uniformi per tutto il territorio nazionale, da Aosta a Trapani. Prevedere, inoltre, che esista una procedura autorizzativa, che sia unica per la stessa tipologia di impianti, significa non solo far bene all'ambiente, ma evitare anche una sorta di *dumping* industriale,

Le Agenzie regionali, dove già esistono eccellenze di grande livello, avranno in questo schema più autonomia, e anche l'ISPRA, in questo disegno, assume un ruolo più importante: non solo di supporto tecnico ai ai Ministeri, ma di perno di un sistema nazionale. All'ISPRA e ai suoi lavoratori va la mia solidarietà. Credo sia importante in questo momento finanziare di più la ricerca e il monitoraggio e in futuro finanziare meno gli interventi di bonifica ambientale, che molte volte sono fatti anche da chi ha provveduto a inquinare. Sicuramente alcuni nodi rimangono irrisolti, lo sappiamo; ogni provvedimento è migliorabile,

Onorevoli colleghi, avverto che è stata chiesta dal senatore Buccarella la dichiarazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 1959, recante l'estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura per il perseguimento di taluni nuovi delitti. Ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, la discussione su tale richiesta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, mercoledì 18 maggio. Seguirà la votazione per alzata di mano. **Interventi su argomenti non iscritti

*(Misto)*. Signora Presidente, lo scorso venerdì, a Livorno, prima del Consiglio comunale che verteva sull'avviso di garanzia al sindaco Nogarin e all'assessore al bilancio per il reato ipotizzato di bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'inchiesta sulla municipalizzata, il consigliere di opposizione Marco Valiani è stato aggredito davanti al palazzo comunale. Sembra - ed è stata presentata denuncia in tale senso - che l'autore dell'aggressione sia il marito di una consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Si tratta di un fatto grave, sia perché dà prova dell'incapacità di una forza politica di mantenere il confronto politico sui binari della democrazia, sia perché non ho letto di alcuna condanna dell'atto da parte di loro rappresentanti locali o nazionali. Richiamo pertanto all'attenzione delle massime autorità istituzionali la situazione di Livorno, che tanto ha dato alla storia di questo Paese, e la punizione oltremodo a cui sono condannati i suoi cittadini che avranno modo, appena gli sarà data la possibilità di votare - se quel sindaco e quella Giunta lo consentiranno - di sanzionarli con il il libero voto. Per quanto ci riguarda, e soprattutto mi riguarda, non è possibile minimizzare quei fatti - ripeto, soprattutto perché non ho sentito sollevarsi alcuna voce di condanna - che costituiscono ben più di un campanello d'allarme di quello che alberga nelle viscere del Movimento 5 Stelle. È già successo in tempi bui, che hanno preceduto l'avvento della nostra Costituzione, che sia stata tollerata per cinico calcolo la violenza dello squadrismo, e abbiamo visto dove il fascismo ci ha portato. Così come allora, permettere questo stato di cose facendo finta di nulla - e per la mia originaria appartenenza ne sento maggiormente la responsabilità - rende complici e non si può né si deve tacere. Ribadisco la mia totale solidarietà a Marco e a quei cittadini che con lui sono opposizione in quel Comune.

Queste le affermazioni molto interessanti di Roberti: legalizzare la vendita di *cannabis* consentirebbe di assestare un duro colpo ai combattenti dello Stato Islamico così come alla criminalità organizzata italiana. La principale strada percorsa dalle partite di *cannabis* passa per Casablanca, in Marocco, raggiunge l'Algeria, la Tunisia e quindi arriva fino a Tobruk, nella Libia orientale. Su tale percorso si trova Sirte, città che rappresenta uno sbocco sul Mediterraneo in mano ai miliziani dell'ISIS. Questi ultimi controllano certamente la via libica. Aggiunge poi Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, che le indagini hanno portato alla luce prove di legami instaurati tra i combattenti islamici e i narcotrafficanti italiani. Un sodalizio, quello tra mafia e Stato Islamico, che consente a quest'ultimo di sfruttare una quota dell'immenso e florido traffico di droga della criminalità organizzata, che vale - secondo le stime dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine - oltre 32 miliardi di euro l'anno (quasi due redditi di cittadinanza). Franco Roberti lo conoscete e penso che lo stimiate. In Parlamento giacciono varie proposte, una, tra l'altro, dell'intergruppo rilanciata dal sottosegretario Della Vedova, che vede la firma di più di 300 parlamentari.

A questo punto dico: o questo Governo e questa maggioranza fondamentalmente non vogliono capire, sono stolti e ignoranti, oppure sono collusi con la mafia. Se questa è una via, un'arma per il contrasto alla mafia, ma ma soprattutto al terrorismo (senza parlare di tutti gli impieghi eccelsi di questa pianta in ambito industriale, medico, sanitario e quant'altro), non legalizzarla significa che probabilmente ci sono degli interessi di questo Governo e di questa maggioranza che vanno contro il Paese e a favore della mafia,

«è inaccettabile che l'orientamento sessuale» determini «offese», discriminazioni o «aggressioni», così come è inaudito che «ciò determini discriminazioni sul lavoro e nelle attività sociali ed economiche». Queste sono alcune delle belle parole che questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mettere per iscritto in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale contro l'omofobia che si celebra il 17 maggio, in particolare in Europa, come ricorrenza ufficiale istituita nel 2004 dalle istituzioni europee. Ed è stato molto utile e bello che oggi, non per la prima volta, il Ministero dell'istruzione abbia voluto inviare a tutte le scuole italiane una circolare in cui invita le scuole a mettere in campo delle azioni concrete per combattere tutte le discriminazioni e, fra queste, anche anche la discriminazione omofobica. Questo naturalmente non significa che nel nostro Paese l'omofobia sia in calo; anzi, proprio in un momento, come è accaduto anche in altri Paesi nelle stesse circostanze, in cui i diritti delle persone omosessuali entrano finalmente a fare parte del corpo legislativo del Paese, entrano nel dibattito pubblico in primo piano, ecco che aumentano anche gli episodi e le recrudescenza omofobiche. D'altra parte, oggi Arcigay, come tutti gli anni, ci ha consegnato un corposo *report* degli atti di omofobia accaduti negli ultimi dodici mesi, che ne elenca 104: sono solo quelli emersi e visibili, solo quelli riportati dai quotidiani del nostro Paese. Fra questi, due omicidi, due suicidi, più tanti casi di omofobia di tipo molto diverso. Voglio solo citarne alcuni perché non si pensi che queste cose non esistano. Vorrei partire da un fatto accaduto il 17 maggio dello scorso anno. Nella Giornata contro l'omofobia, di fronte a un gruppo che manifestava per il contrasto all'omofobia, un gelataio ha esposto un grande cartello in cui c'era scritto «genitori, tenete lontani i vostri figli dai gay»: un gesto simbolico in quella giornata. Ma ci sono tante cose molto più gravi, come il caso di quel turista olandese di quarantun anni aggredito insulti e percosse sul lungomare di Catania; come il caso di quel bambino di pochi anni che nella propria scuola è stato ripetutamente insultato finché la madre ha denunciato pubblicamente il fatto; fino al caso casa e ai tantissimi - come dicevo più di cento - casi accaduti lo scorso anno. Il Parlamento deve per questo fare la sua parte. Noi oggi abbiamo chiesto, come Gruppo del Partito Democratico, in Commissione giustizia del Senato che si riprenda l'*iter* della legge contro l'omofobia, impropriamente all'esame della proposta di legge sull'istituzione, anche da parte del Parlamento italiano, della Giornata nazionale contro l'omofobia. Oggi abbiamo depositato, insieme a tanti altri senatori, un disegno di legge contro le cosiddette terapie riparative, quegli odiosi interventi di pseudo-guarigione dei ragazzi e delle ragazze omosessuali dalla loro identità, sessualità e personalità. Mi auguro che, non solo attraverso gli atti formali che ho citato, ma anche attraverso atti normativi, questo Parlamento voglia dare un segno concreto per l'abbattimento di quell'altissimo livello di omofobia ancora presente nel nostro Paese. *(Applausi *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, intervengo brevemente per esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza ad Alessandro Marcelli, attivista del Movimento 5 Stelle di Tagliacozzo, vittima, mentre stava lavorando nella sua lavanderia, di un ignobile atto di aggressione compiuto da tre uomini incappucciati, che nascondevano il loro volto. Esprimo la solidarietà di tutto il Gruppo per Marcelli, che ha sporto ovviamente denuncia e le indagini sono in corso. Tra le ipotesi che vengono fatte dagli inquirenti c'è quella che l'aggressione, tra l'altro verificatasi nel giorno in cui nel suo negozio avrebbe dovuto svolgersi la riunione del *meetup* locale, sia riconducibile al suo impegno politico con il Movimento 5 Stelle e che sia un'aggressione che possa riguardare la lista che si presenterà alle prossime elezioni amministrative nella cittadina abruzzese

se la pista politica venisse confermata. Sappiamo che possiamo essere spesso scomodi per qualcuno, ma è assolutamente inaccettabile che si usi la violenza fisica o psicologica per intimidire. L'episodio accaduto si aggiunge tristemente ad una lunga serie di queste azioni spesso subite da persone del Movimento, come la casa del sindaco di Pietraperzia

le soluzioni ai problemi le troveranno insieme e non ci sarà spazio per chi non ha adeguati argomenti e usa la violenza e gli atteggiamenti di bullismo e prevaricazione solo per intimidire.